Grazie

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

A mio avviso, le aperture vanno fatte con molta cautela. Ieri sentivo parlare in quest'Aula delle RSA. Per conoscenza personale di situazioni, penso sia il luogo più delicato ove bisogna procedere con santa pazienza sia per gli ospiti che per i parenti. buona cosa avere fissato un calendario per le aperture; speriamo che, con i dati favorevoli, la situazione possa addirittura migliorare. Il discorso sulle aperture mi offre lo spunto per una breve digressione.

L'opinione pubblica si è schierata dalla parte di Abele, dalla sua parte, perché l'orefice siamo noi, pur provando pietà e compassione per i morti. La legge sta facendo il suo corso: avviso di garanzia come atto dovuto, indagini molto approfondite nell'immediato e l'autopsia che - pare da fonti giornalistiche - ha stabilito che i banditi sono stati colpiti in faccia e non in fuga. è un attimo, dura pochi secondi, un minuto al massimo; il cervello, l'istinto, la paura, il proprio passato che si intravede in un attimo. Vorrei che risuonasse in quest'Aula il nome di Mario Roggero perché è uno di noi, un italiano che lavora, che vorrebbe lavorare tranquillo e sicuro, che ha fatto e che fa l'Italia. Gli auguro un *iter* giudiziario che non sia un calvario; auguro a lui e alla famiglia di avere la forza di ripartire, con la solidarietà e l'amicizia di tanti, della maggioranza silenziosa, in rappresentanza dei valori forti che fanno la nostra società. Il decreto-legge n. 41: essere maggioranza. Credo che si possa ancora registrare all'interno dei partiti, del vasto schieramento che appoggia il Governo, il fatto di classificarsi, noi e voi - quelli che erano maggioranza prima e quelli che si sono aggiunti ora - secondo un discorso di parità. Penso che gli emendamenti soprattutto di tipo ordinamentale possano essere discussi, e ce ne sono di importanti (quelli ordinamentali normalmente non comportano Altrimenti questa Camera, la Camera alta, non ha l'opportunità di discutere e di decidere nulla, perché i disegni di legge, data l'incombenza dei lavori per motivi che non conosco, ma che comunque non mi piacciono, non vengono discussi. Ad esempio, io avevo presentato un emendamento sui cosiddetti sovraspessori nelle costruzioni, per i casi in cui vi sia una nuova costruzione, per migliorare la prestazione energetica oppure degli interventi di riqualificazione ai fini energetici degli edifici esistenti, affinché si possa derogare all'aumento dei volumi, secondo secondo un sistema di calcolo, rispetto ai muri e alle solette. Non è banale, perché da questo emendamento, che spero di poter riproporre e discutere col Ministero competente e di far sottoscrivere da tanti colleghi, possono derivare benefici effetti sul famoso

È vero che è cambiato il sistema di calcolo, ma questi contributi non bastano mai. Purtroppo, per la ripartenza serviranno in misura maggiore: di questo siamo tutti o quasi tutti coscienti. Bisognerebbe approfittare di questo momento per studiare e normare le trasformazioni della società, le trasformazioni del lavoro, regole per stare dentro. Io penso che tanti ristoranti e bar, purtroppo, non riapriranno, ma perché alcuni non hanno neanche i requisiti rispetto alla pandemia e a ciò che ne deriva e ne deriverà. Chi starà fuori dovrà essere oggetto di *welfare* oppure di nuovo lavoro, che può derivare dal PNRR, se ci crediamo veramente tutti e se normiamo e stabiliamo tutto quello che c'è da modificare: secondo le prescrizioni dell'Europa, sì, ma a nostra utilità e a uso dell'Italia.

dal MEF, in data 6 ottobre 2020, che dice che il magazzino fiscale, del quale qualcuno qui dentro si riempie la bocca, che era di 986 miliardi, in realtà è di 74 miliardi.

dei quali bisogna prendere atto con un provvedimento. Questo perché non esistono: i 74 miliardi vanno divisi per due e derivano, per la maggior parte, da crediti dello Stato o di altri enti e qualcosa dall'INPS.

per 1,928 miliardi - sono i fondi meglio stanziati - e 2,8 miliardi per comprare nuovi vaccini. I vaccini vanno comprati ad ogni prezzo: lo dico per la terza volta in quest'Aula. 500.000 vaccini al giorno è un traguardo giusto, ma è un punto di partenza. Sulla base dei dati, stante il fatto che bisogna essere vaccinati due volte, occorrono 200 giorni totali per vaccinare tutti, meno i già vaccinati. Dopodiché, bisogna ripartire.

confido che il Governo possa ottenerla e possa stanziare delle

Finalmente il Parlamento ha riacquisito un ruolo centrale nel processo legislativo. Il provvedimento eroga lo scostamento da 32 miliardi di euro, votato a gennaio dal Parlamento, per far fronte alle esigenze del protrarsi della pandemia oltre il periodo di Natale e indennizzare le attività produttive danneggiate a dicembre e gennaio scorsi. Certo, ormai siamo a maggio e ancora non siamo tornati alla normalità, né alla riapertura totale delle nostre attività questo ci ha costretti a un ulteriore scostamento di bilancio per ulteriori 40 miliardi di euro che saranno impiegati per il prossimo decreto Siamo consapevoli che il miglior sostegno che possiamo dare è quello di far tornare alla normalità il Paese al più presto. Lo sforzo del generale Figliuolo di procedere velocemente nella campagna vaccinale è sicuramente la strada giusta per consentire le riaperture e far così ripartire l'Italia in maniera spedita verso la ripresa economica.

Vorrei parlare di montagna, che è un tema a me caro per le mie origini e per la mia appartenenza a un territorio bello, che, proprio per la sua caratteristica morfologica, vede le attività economiche basarsi quasi esclusivamente sul turismo, mentre le rimanenti godono, a ricaduta, dei benefici che questo settore comporta. Non ricordo un inverno così nervoso da quando ero bambina, ma soprattutto non ricordo un silenzio così assordante come quello che la passata stagione invernale ha riservato alle località turistiche di montagna. Qualcuno in principio ha cercato di banalizzare la mancata stagione invernale dicendo: è solo una sciata. Cosa più sbagliata non si poteva dire perché chi vive in montagna sa che il lavoro di una stagione invernale significa, in parole povere, poter fare la spesa, pagare il riscaldamento, le tasse universitarie, l'affitto di casa e così via. Insomma, Sulla base dei dati dell'Osservatorio italiano del turismo montano, nell'inverno 2018-2019 il comparto, nelle sole 61 principali stazioni sciistiche italiane, ha riportato un fatturato pari a 10.409 milioni di euro. I lavoratori del comparto sono stimati in circa 75.000 unità. Pertanto, il fatturato perso è stato veramente ingente, soprattutto per quelle attività (impianti sciistici, maestri di sci, noleggio di attrezzature invernali) che purtroppo hanno il loro introito solo nei mesi invernali. Oltre al mancato incasso o stipendio, si deve tener conto dei costi fissi, spesso alti. Consideriamo che le temperature sotto lo zero comportano la

La notizia del *premier* Draghi di un *green pass* nazionale ci dà grandi speranze e soprattutto ci mette alla pari con i nostri *competitor* europei. Almeno non ci saranno corsie preferenziali verso le località estere, così il prodotto turistico italiano può concorrere ad attrarre i turisti stranieri. Questo messaggio di fiducia dà sollievo ad un comparto che necessita di poter programmare la ripartenza ed avere la certezza di poter fare almeno una buona stagione estiva. sua nascita, questo nuovo Governo ha esordito bene, con l'istituzione del Ministero del turismo, e voglio ringraziare il ministro Garavaglia per l'impegno e l'attenzione che dimostra per le diverse specificità del turismo che l'Italia offre. L'articolo 2 del decreto sostegni è interamente dedicato a misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, con un fondo di 700 milioni così ripartito: 430 milioni per gli impianti di risalita, 40 milioni per i maestri di sci e scuole di sci e i restanti 230 saranno divisi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e destinate alle imprese turistiche operanti nei comprensori sciistici. È stato inoltre approvato in Commissione un ordine del giorno per incrementare il fondo di 100 milioni nel prossimo decreto sostegni *bis.* Grazie anche agli emendamenti della Lega, sono state inserite una serie di misure immediate e concrete per dare ossigeno ai nostri commercianti, per dare un aiuto vero alle categorie più colpite dalla crisi: lo *stop* al pagamento della rata dell'IMU di giugno per i beneficiari dei ristori; la sospensione del del pagamento della TOSAP e della COSAP; l'esenzione del pagamento del canone RAI per bar, pub e ristoranti; il rinvio al 30 settembre del pagamento dell'IRAP da parte delle imprese. Tutto questo, però, ovviamente non è sufficiente, non basta e per questo lavoriamo perché nel prossimo decreto sostegni siano previste ulteriori azioni e misure a favore delle imprese. Servono ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA e di imprese che hanno

c) misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese (PMI) e a prorogare fino al 31 dicembre 2021, la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti; Bisogna stanziare adeguate risorse in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tari da parte delle imprese. Bisogna prorogare l'indennità a favore dei lavoratori stagionali di vari comparti (agricoltura, turismo e spettacolo). Questa crisi ha portato con sé tanti problemi, si contano purtroppo già quasi un milione di posti di lavoro persi e c'è ancora il blocco dei licenziamenti. Far ripartire l'economia significa rigenerare posti di lavoro, dare sicurezza alle famiglie che in questo periodo, oltre al fattore economico, hanno dovuto fare i conti con le difficoltà insorte dalle restrizioni, con ricadute dannose anche sotto l'aspetto psicologico. Pensiamo alle difficoltà a cui bambini e adolescenti hanno dovuto adattarsi, che sono state molteplici: la chiusura delle scuole, la sospensione delle attività sportive, sociali e ricreative, le ore passate davanti al PC, dato loro la visione di una società fatta di isolamento, che sicuramente ha creato forti disagi anche per tanti nostri giovani che devono affacciarsi al mondo del lavoro e si ritrovano sfiduciati. Abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le azioni che preservino la qualità della nostra vita. Abbiamo il dovere di ringraziare chi è in prima linea dall'inizio della pandemia e mi riferisco ai medici, agli operatori sanitari che ancora oggi sono impegnati nella campagna vaccinale e ai tanti volontari. Questo impegno profuso ci permetterà di ripartire e di vedere le nostre piazze, i pubblici esercizi e le località turistiche tornare a vivere. In questi giorni finalmente ci sono state le prime riaperture di bar e ristoranti, per ora solo all'aperto, cosa che per le attività in alcune località, come quelle montane, è molto difficoltosa, viste le temperature, pertanto l'obiettivo resta dare la possibilità di lavorare in sicurezza a chi è ancora fermo e su questo dobbiamo impegnarci. La voce della Lega, che all'interno del Governo lavora per dare uno spiraglio di luce dopo questo periodo così difficile, ci rende fiduciosi che gli obiettivi che ci siamo prefissati possano e debbano essere raggiunti per una ripresa economica forte, che concorra al benessere omogeneo del Paese senza lasciare nessuno indietro e tenendo sempre puntato lo sguardo sulla tutela della salute. Qualcuno ha definito la pandemia come una guerra contro un nemico invisibile. Mi ricordo che quando ero bambina mia nonna mi raccontava tutte le difficoltà che aveva affrontato durante la guerra, compresa la paura, la fame e il terrore di perdere i propri cari. Da loro, dai nostri nonni, dovremmo prendere esempio, non arrenderci e affrontare le difficoltà con determinazione e con il e con il coraggio di esporci in prima persona per trovare le soluzioni migliori. Per questo sono orgogliosa della scelta di Matteo Salvini di far parte del Governo perché metterci la faccia e provare a portare le soluzioni giuste, assumendosene la responsabilità, non è cosa da tutti.

un percorso mai interrotto e fatto di aiuti economici e misure emergenziali, indispensabili per fronteggiare l'emergenza dovuta alla pandemia. Le risorse messe in campo con il provvedimento al a 32 miliardi di euro e sono il frutto dello scostamento di bilancio votato a gennaio con il Governo Conte-*bis*, che è stato fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle. Fin dal primo momento infatti il MoVimento 5 Stelle si è battuto fermamente per ottenere risorse dall'Europa e per far sì che fossero utilizzate nel migliore dei modi. Ci rendiamo conto che quanto fatto non è ancora abbastanza e siamo consapevoli delle difficoltà estreme che tutti stiamo fronteggiando, ma siamo convinti che è ancora tanto quello che riusciremo a realizzare. Da sempre siamo accanto ai cittadini, alle famiglie e agli imprenditori perché siamo nati dal basso della società civile, come forza propulsiva del cambiamento e quel cambiamento lo abbiamo inciso nel nostro DNA. Dalle piazze italiane urlavamo che nessuno deve rimanere indietro; possiamo essere fieri nel dire che non è rimasto solo uno *slogan*, ma che è la rotta costante delle nostre scelte in Parlamento. L'emergenza ha permesso di adottare interventi senza precedenti nel dare ossigeno alla nostra economia, messa a dura prova dalla pandemia, e nel dare conforto materiale ai cittadini in difficoltà. reso possibile riconsiderare le priorità e fare scelte coraggiose per mettere liquidità e sostenere imprese e famiglie. Non si tratta certo di assistenzialismo, ma di un sostegno indispensabile per rafforzare le difese organiche della nostra società che sta fronteggiando la crisi più profonda dei nostri tempi. Misure come il reddito di cittadinanza che, ad esempio, sarebbero state impensabili solo pochi anni fa, vengono oggi non solo confermate dal Governo Draghi, ma implementate con il decreto-legge sostegni. Se oggi il sistema tiene, è anche per merito del reddito di cittadinanza, che ha permesso di supportare migliaia di famiglie in difficoltà. Ne è prova Ne è prova la continuità delle scelte dell'attuale Esecutivo con il precedente, che ha confermato anche gli incarichi di collaborazione dei *navigator* fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica nei centri per l'impiego. Per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, la decisione di abbandonare la classificazione per il codice Ateco è una presa di coscienza della possibilità di migliorare i provvedimenti passati. Si è scelto il criterio del calo di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019, senza limitazioni a categorie professionali, con una progressività del contributo a fondo perduto che è maggiore tanto più piccola è l'azienda, nella consapevolezza che le medie e piccole imprese sono quelle più a rischio in questo momento. Per salvaguardare le attività più colpite dalle restrizioni adottate per contenere i contagi, sono state pensate ulteriori misure economiche; ad esempio, sono stati istituiti nuovi fondi a sostegno del turismo invernale e sono state previste indennità per i lavoratori stagionali, per i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali e anche per i lavoratori dello spettacolo e dello sport che, a causa della pandemia, hanno cessato e sospeso la loro attività. Inoltre, come componente della Commissione parlamentare

come alberghi, case vacanze, *bed and breakfast*, villaggi turistici e campeggi, nonché i bar e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui si somministrano e consumano bevande, a cui si aggiungono tutti gli enti del terzo settore. Per coloro i quali avessero già provveduto al pagamento del canone speciale è stato previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione corrispondente all'importo versato. Da tempo mi occupo personalmente del tema del canone RAI e a tal proposito ho presentato già nel 2019 un disegno di legge per modificarne la disciplina. Inoltre, a seguito della pandemia e delle gravi perdite subite dalle attività che pagano il canone speciale, ho depositato anche un'interrogazione scritta al Ministero dello sviluppo economico affinché si occupasse del problema. Oggi, grazie al decreto-legge sostegni, possiamo ritenerci soddisfatti. Sono infatti convinta che tale misura sia un concreto aiuto per queste attività; ogni piccolo passo è un passo verso la ripresa, la strada è lunga, ma possiamo garantirvi che non ci fermeremo. Insieme, con la responsabilità politica che ci tiene saldi a questo Esecutivo, sono convinta che riusciremo ad uscire dall'emergenza

dal cui nome stesso si evince l'intento del Governo di sostenere, attraverso i vari articoli, un Paese che ancora oggi sta lottando contro la pandemia, anche se i dati dei contagi pian piano sembrano apparire confortanti rispetto ai mesi scorsi. L'effetto è dovuto sicuramente alla campagna vaccinale che sta incentivandosi,

Signor Presidente, faccio un appello per i nostri connazionali italiani: penso a quella coppia che è andata ad adottare una bambina in India, affinché si faccia tutto il più possibile per farli rientrare in Italia. Lei teme per la sua salute, quindi faccio questa richiesta prima di tutto il resto.

ampliare una volta per tutte la possibilità di vaccinare a coloro che possono farlo e nei luoghi dove ciò si può fare, per evitare di incorrere sempre in tutte quelle lotte fra professionisti che non ci devono essere. *(Applausi)*. Quindi facciamolo una volta per tutte, credo che sia importantissimo.

ha senso. Se queste persone finalmente ricoprono il ruolo a loro dovuto, lo devono fare per sempre e non solo relativamente all'emergenza Covid; questo è un altro dato importante.

Questa è un'altra cosa importantissima; è inutile che vi dica quanto è grande il disagio e il malessere psicologico che i bambini, gli adolescenti e di conseguenza le loro famiglie stanno sopportando. Ho sentito prima nella per l'infanzia e l'adolescenza che ci sono dei casi incredibili di ragazzi che usano addirittura sostanze stupefacenti per passare questo periodo, che purtroppo è gramo un po' per tutti, ma soprattutto per i nostri ragazzi. Credo che questo, insieme all'approvazione

dal rafforzamento della medicina del territorio, ed è quello che noi troviamo nella missione 6 del PNRR, di cui attendiamo a breve l'approvazione della Commissione europea e la stesura di progetti concreti da condividere con tutti gli attori interessati, *in primis* con il Parlamento. *(Applausi)*. Grazie Signor Presidente, questo decreto-legge è un vero e proprio spartiacque che segna la differenza non solo tra due Governi, ma anche tra modi opposti di rispondere alla crisi. Siamo passati dal rincorrere gli effetti del Covid a finalmente governarli. Questo Governo ha impresso quel cambio di passo che chiedevamo e che era necessario per portare il Paese fuori dalla pandemia. Non voglio soffermarmi su aspetti economici di cui hanno ampiamente parlato i miei colleghi, bensì sui due aspetti sul fronte sanitario di cui sono particolarmente soddisfatta. Sostenere significa recuperare il tempo perso, vorrei dire sprecato nelle mancate cure. Il Covid non ha soltanto causato 122.000 vittime dirette, ma ha ucciso donne e uomini che avevano altre patologie e che non hanno potuto curarsi. Oggi rimediamo a un errore pericoloso. Attraverso un emendamento abbiamo chiesto che pazienti oncologici in *follow up* venissero inseriti tra le categorie vulnerabili. Parliamo di persone che hanno avuto una diagnosi di tumore e che hanno affrontato trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni. Grazie a questa modifica, i malati più esposti al rischio di contrarre il Covid potranno effettuare il vaccino con le stesse modalità e la stessa tempistica con la quale possono accedervi tutte le altre persone considerate fragili. Fino ad ora, infatti, queste persone, nonostante la loro evidente fragilità, non godevano di alcuna priorità. Considero per questo il parere del Governo e la decisione della maggioranza di inserire questo emendamento all'interno del decreto un gesto di grande attenzione nei loro confronti.

potranno inoculare i vaccini contro il Covid. Averle abilitate alla somministrazione del vaccino è un atto di buon senso, di razionalità, un gesto di considerazione nei confronti di 2.700 donne generose, ma soprattutto un'ulteriore spinta per la campagna vaccinale. Come segnalava la Croce Rossa, che sabato celebra la sua festa, le crocerossine sono formate attraverso un corso di due anni, al termine del quale possono anche effettuare iniezioni intramuscolo in presenza del medico. Questo personale, già attualmente impegnato presso gli *hub* vaccinali, darà il suo contributo allo sforzo corale che sta facendo l'Italia in tutte le sue articolazioni per raggiungere l'immunità di gregge che ci renderà finalmente liberi. *(Applausi)*. Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile. ancora lontani dall'avere il Paese che ci chiedono gli italiani, quello che serve alle aziende per prosperare o almeno per tornare a crescere: un'Italia sicura e che garantisca a tutti la salute e il benessere. discussione, contenente queste misure positive, sono la ragione per cui abbiamo voluto dare il nostro contributo al Governo Draghi e vogliamo continuare a darlo. Un piano vaccinale efficiente che funziona e procede in modo spedito e che, grazie anche alle modifiche introdotte in questo decreto-legge, correrà ancora più velocemente è la migliore risposta al terrorismo psicologico esercitato dai no vax, i quali non capiscono che i vaccini sono la soluzione al Covid e non la causa. *(Applausi)*. È la migliore risposta a chi, rifiutando di immunizzarsi, mette a rischio non solo la propria vita, ma soprattutto quella degli altri; è la migliore risposta della scienza all'ignoranza. Sono queste le tante risposte che stiamo dando al Paese, a tutti gli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori che hanno voglia di ripartire e che, per farlo, hanno bisogno che la sicurezza sanitaria sia garantita. Lo stiamo facendo e con questo decreto, come modificato qui in Senato, la strada per tornare alla normalità si è accorciata ed è diventata meno tortuosa.

ad andare nel verso giusto. È il primo importante provvedimento di questo Governo, che ha emanato un decreto-legge subito esecutivo e il Senato e i senatori tutti hanno cercato di dare il loro apporto migliorativo. quindi i due relatori, i senatori Roberta Toffanin e Daniele Manca, per il lavoro di mediazione svolto al fine di trovare un accordo tra le forze di maggioranza e anche di minoranza.

ma è sbagliato non avere qualche ora in più per approfondire e non avere il tempo per coinvolgere i colleghi nelle scelte. È sbagliato non avere a disposizione i testi e procedere ugualmente alle votazioni. È sbagliato, colleghi, ridursi sempre a lavorare di notte. Ho sempre sostenuto - e lo ribadisco qui in Aula - che il lavoro fatto di fretta e di notte rischia di essere viziato da errori. Non parliamo, poi, di alcuni tentativi di propinare emendamenti non concordati; forse è un errore, ma mi domando se non sia una scorrettezza. Comunque andiamo avanti così e cerchiamo di non fare scorrettezze.

di questo nuovo Governo andrà a finanziare il secondo decreto sostegni, che vedrà la luce nei prossimi giorni. Ebbene, in pieno accordo tra i Gruppi, abbiamo individuato alcune tematiche onerose, da gestire con emendamenti comuni, e altre molto onerose e impossibili da trattare nel primo importanti e da rimandare al decreto sostegni-*bis*, per le quali abbiamo quindi concordato un ordine del giorno. Per quanto riguarda il primo articolo, sul fondo perduto, abbiamo ottenuto di superare l'intricata e inefficiente logica dei codici Ateco, sostenendo, seppur nei limiti dello stanziamento iniziale, tutte le attività che hanno subito una perdita di fatturato superiore al 30 per cento. A tal proposito, con un nostro emendamento, si è stabilita l'impignorabilità del contributo a fondo perduto. Nell'ordine del giorno si è chiesto inoltre l'impegno del Governo a prevedere ulteriori contributi a fondo perduto nel prossimo decreto ristori. Si è altresì chiesto un impegno con particolare riguardo ai costi fissi, ai canoni di locazione su immobili ad uso non abitativo, agli affitti d'azienda e alla quota fissa delle bollette elettriche. A proposito di affitti, si è iniziato in questo provvedimento, con emendamenti e di altri Gruppi, a dare un primo segnale di attenzione ai proprietari di immobili ad uso abitativo (mentre per quelli commerciali si è rimandato al decreto per esentarli dal pagamento dell'Irpef su canoni di locazione non percepiti. Si è inoltre agito per bloccare gli sfratti, almeno quelli avviati prima della pandemia.

Si è, poi, agito in diversi altri settori. La montagna è un tema che mi sta particolarmente a cuore, come piemontese, e di cui ha già ben parlato la collega Testor. Con un ottimo lavoro del ministro Garavaglia in Conferenza Stato-Regioni, abbiamo stabilito in questo provvedimento i criteri di riparto, con l'impegno sul decreto sostegni-*bis* di aumentare il fondo dedicato alla montagna di 100 milioni Si è agito sull'esenzione TOSAP e COSAP per le attività costrette alla chiusura, demandando al decreto sostegni-*bis*, con un impegno del Governo, l'esonero del pagamento della Tari

di convogliare ulteriori 50 milioni di euro per dare un sostegno alle società sportive dilettantistiche, lasciate fuori dai precedenti provvedimenti. La Lega, poi, ha dimostrato un'attenzione particolare per la disabilità, con l'instancabile lavoro del del ministro Erika Stefani, e, come ha ben evidenziato ieri il collega Augussori, sono stati portati avanti emendamenti importanti. Mi riferisco alla finalizzazione del fondo per le disabilità, alle risorse *pro* ciechi e alla battaglia, su cui tanto ha puntato il senatore Salvini, insieme a tutti noi della Lega, per il riconoscimento della lingua dei segni. Signor Presidente, questa è soltanto una parte delle misure che abbiamo portato avanti. con le risorse disponibili, abbiamo cercato, per quanto possibile, di sostenere la nostra economia, le nostre attività costrette alla chiusura forzata, nella consapevolezza che il miglior sostegno è dare alle nostre attività l'opportunità di lavorare, di riaprire, di tornare alla normalità, superando quindi la logica del coprifuoco e delle chiusure. *(Applausi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in quest'Aula per manifestare la mia soddisfazione in merito a una serie di provvedimenti che siamo riusciti ad introdurre in questo decreto sostegni. sostegni. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre operato, in questo periodo di pandemia, in maniera molto razionale da un lato, e in maniera molto responsabile dall'altro.

soprattutto nel periodo iniziale, in maniera emergenziale; abbiamo cercato di rendere rapidi i processi amministrativi in un Paese in cui, in realtà, tutti i processi amministrativi informatici

ci sono anche delle attività storico-culturali italiane, ad esempio quella del commercio dei mercati, degli ambulanti. Siamo molto soddisfatti di aver sostenuto la durata e la proroga delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, proprio al fine di garantire la continuità dell'attività a sostegno di questo settore nell'attuale quadro emergenziale. Un altro importante obiettivo raggiunto, del quale siamo veramente contenti, è quello di aver ampliato e quindi sostenuto anche il fondo per i fieristi.

le possibilità di operare, anche perché abbiamo ormai la certezza che in luoghi aperti il virus si trasferisce in maniera molto meno rapida. Sarebbe quindi opportuno, con tutte le sicurezze, riaprire anche

infortuni sul lavoro), che da tempo lavora su casistiche similari per altre tipologie di problematiche collegate ai virus.

Nel decreto sostegni viene incrementato, nella misura di un miliardo e mezzo, la dotazione per il 2021 del Fondo per l'esonero del versamento dei contributi dovuti da lavoratori autonomi e professionisti.

Un'altra particolarità che dà una boccata di respiro è la riduzione della spesa dei consumi elettrici per uso non domestico,

C'è stata proprio la volontà di predisporre nel decreto sostegni-*bis* un'altra serie di provvedimenti. l'azzeramento e l'esonero della tassa sui rifiuti (Tari). Forniremo ai Comuni i fondi necessari affinché le attività economiche possano azzerare anche questa tassa che in questo periodo di pandemia, con le chiusure, è veramente ingiusta. Un'altra cosa su cui sarebbe opportuno, a mio avviso, porre una certa attenzione è l'esonero dal canone RAI. Per questo ringrazio la collega Felicia Gaudiano e il collega Sergio Vaccaro, che hanno voluto fortemente questo esonero dal canone RAI a favore delle strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande. Ancora una volta interveniamo per piccola e media impresa. Un'altra particolarità che abbiamo sostenuto sempre con energia, forza e anche visione, sempre sempre a favore della piccola e media impresa, è l'esonero dal canone per l'occupazione del suolo pubblico che, questa in questo periodo di pandemia, con l'obbligo delle chiusure, veramente risulta una tassa insopportabilmente ingiusta. Un'altra tematica sono le *startup*, per cui devo rilevare il grande impegno del MoVimento, che ha a cuore sempre lo sviluppo della capacità imprenditoriale del singolo individuo al fine di far emergere le potenzialità che possono concorrere al progresso del nostro Paese. Per tale ragione è stato introdotto il contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, è iniziata nel 2019, in un periodo veramente particolare. dobbiamo essere rapidi nell'approvare e credo che ci abbiamo messo tutto l'impegno. Ringrazio, pertanto, tutti i colleghi delle Commissioni che hanno avuto la capacità di interagire con le minoranze per portare in maniera rapida il provvedimento al Paese, ma ricordiamo di essere altrettanto rapidi con il decreto sostegni-*bis* perché ci sono tantissime altre piccole e medie imprese che stanno soffrendo e hanno bisogno del nostro sostegno.

Questo non ci pare dal contenuto del decreto-legge sostegni. Oggi ci sarebbe invece piaciuto conoscere dal Governo una *timetable* sulle aperture nella nostra Nazione.

un'ennesima distribuzione a pioggia, che certamente non servirà né per rilanciare la nostra economia, né per aumentare i consumi degli italiani.

secondo voi chi potrebbe mai prenotare le vacanze nella nostra Nazione, sapendo che alle 10 di sera deve stare chiuso in casa o in albergo? La comunicazione è importante! Non riesco a capire come non siate preoccupati del lavoro, dei lavoratori e della perdita di lavoro che ci sarà, un secondo dopo la fine del blocco dei licenziamenti. Voi invece fate orecchie da mercante!

mese. Pensate veramente di aiutare le imprese dando il sostegno su un mese di fatturato? Nella vita faccio l'imprenditore, ma noi guardiamo all'andamento del fatturato di un anno.

che parte di questa maggioranza aveva stanziato 460 milioni di euro per i banchi a rotelle, che oggi giacciono nei magazzini. Come vi sentite quando incontrate i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori? Come fate a non abbassare il vostro sguardo, dopo che elargite quella che si potrebbe definire un'elemosina o una mancetta?

che si intravede in questo decreto-legge sostegni è che riconoscete il vostro errore per quanto riguarda i vaccini, perché passate da 400 milioni

con questo provvedimento arriviamo a dare ulteriori risposte ai numerosi bisogni che famiglie e imprese hanno manifestato rispetto alle restrizioni che siamo stati costretti ad attuare per via della pandemia. Tutti noi, però, ci auguriamo che questo decreto-legge e il prossimo già istruito siano ormai tra gli ultimi provvedimenti straordinari ed emergenziali, che portano ad attuare misure con risorse ingenti per dare sostegni e aiuti straordinari. Questo perché la speranza è che l'implementazione del piano vaccinale possa portare a una progressiva normalità anche il nostro Paese, permettendo così allo Stato di avviare l'attuazione degli importanti investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal fondo complementare, in modo tale da poter vedere finalmente crescere anche nel nostro Paese l'occupazione, oltre che il Paese stesso in tutte le sue componenti.

un richiamo costante ad investire e a vigilare continuamente sulle misure di sicurezza lavorative. Queste morti, che sembrano emergere da una costante oscurità, nonostante dati drammatici, ci devono far riflettere perché, Presidente, Luana D'Orazio è morta come in una filanda dell'Ottocento e Christian Martinelli è morto come in un opificio del Novecento. Fatti questi ci devono scuotere, ma ci devono anche indurre a far sì che gli investimenti importanti che lo Stato attuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni pongano il tema della sicurezza

il Parlamento ha avuto un ruolo limitato per quanto riguarda le risorse a disposizione; tuttavia, ha avuto un ruolo significativo nella determinazione delle misure e dei provvedimenti. Anche grazie all'impegno del Gruppo PD, PD, assistiamo a un'importante riduzione dei costi fissi soprattutto per i pubblici esercizi e per gli operatori del turismo. In questo modo si è dato ascolto a tante richieste degli *stakeholder*. Sappiamo che questa deve essere ancora la strada da attuare con l'utilizzo dell'ulteriore scostamento già deliberato dal Parlamento di 40 miliardi, che vedrà l'impiego parziale di quelle risorse nel provvedimento atteso che il Governo sta per varare.

che sono una cellula vitale per il nostro Paese perché sono stati e sono protagonisti nell'aiuto alle famiglie e alle imprese. Credo che si dovrà necessariamente andare nella direzione di coprire completamente, almeno con 600 milioni di euro, lo scoperto che i Comuni registreranno sulla Tari, perché se vogliamo abbattere come costo fisso per le imprese una tassa come quella sui rifiuti dovremo garantire al Comune la piena copertura delle risorse, altrimenti il meccanismo vedrà scaricare sulle famiglie

c'è, poi, un'importante misura legata alla solidarietà alimentare. Abbiamo visto come abbia funzionato bene nei mesi passati dello scorso anno il bonus spesa che è stato riconosciuto alle famiglie bisognose attraverso i Comuni. Questa misura non solo deve essere implementata, ma deve essere resa più flessibile, lasciando ai Comuni le risorse necessarie per dare risposte sulle esigenze di spesa, ma anche sulle coperture di bollette o di affitti per quelle famiglie che i Comuni stessi sanno essere in condizioni di difficoltà. I Comuni sono la sentinella sul territorio per conto dello Stato. Conoscono i propri cittadini, conoscono i bisogni che essi registrano e, quindi, sono i migliori organismi dello Stato, titolati a indicare indicare dove destinare le risorse. L'appello che faccio al Governo, quindi, non è solo quello di destinare le risorse a copertura di queste misure per i Comuni, ma anche quello di rendere flessibile l'utilizzo di tali risorse in funzione delle capacità che ogni singolo Comune sa mettere in campo per riconoscere i bisogni delle famiglie e delle imprese. i Comuni sono stati in prima linea nella gestione della pandemia. Sono stati essenziali e continuano ad essere essenziali nella implementazione del piano vaccinale, perché hanno saputo mettere in campo e coordinare i volontari che assistono i numerosi centri vaccinali e gli operatori sanitari. Saranno protagonisti della ripartenza con gli investimenti previsti dal PNRR. È necessario un patto, lo chiedo al Governo: un patto tra Stato e Comuni per le ragioni che ho indicato, per il ruolo che esercitano i Comuni. i Comuni. Sarà necessario che il Governo affidi responsabilità e risorse, ma anche adeguata autonomia ai Comuni, per delle risposte migliori nei confronti delle famiglie e delle imprese.

senatrice Toffanin e il senatore Manca, per l'ottimo lavoro che hanno svolto, di sintesi e di attenzione ai lavori della Commissione, i due Presidenti di Commissione, senatori Pesco

Personalmente, io di notte faccio fatica a stare sveglio e, per questo, auspico per il futuro che non ci siano notturne. Al di là di questo, venendo al decreto sostegni,

Praticamente, è un decreto sostegno, nel senso che sosteniamo perché vogliamo far lavorare le nostre imprese, vogliamo far lavorare i nostri piccoli e medi imprenditori e vogliamo far ritornare il Paese alla normalità

fermi da un anno e mezzo e il sostegno, per quanto importante possa essere, sicuramente non risolve i problemi. Quindi, bisogna dare fiato e aiuto, dare una boccata di ossigeno, per permettere che, alla riapertura, ci sia la ripartenza. Vedete, colleghi, non si può riaprire e non ha senso riaprire se poi non si riparte. Il nostro sistema produttivo è in difficoltà, i dati stanno testimoniando, e servono funzioni innovative. Chi ha idee nuove è il momento che le tiri fuori e le metta a disposizione del Paese. Il nostro partito, all'appello del Presidente della Repubblica di abbandonare le maglie della propria squadra e di indossare la maglia della Nazionale, ha risposto immediatamente, senza indugio, perché qui è in gioco il Paese. Qui non si tratta di essere

Il presidente Draghi è una garanzia per noi, è una garanzia che non possiamo permetterci di sprecare. Pertanto, anche le legittime osservazioni e critiche devono tornare nell'ambito di un'autorevolezza che nel presidente Draghi trova la sua massima espressione. Lo abbiamo dimostrato: il primo PNRR ci è stato mandato sostanzialmente a casa dicendo che era poco più che carta straccia.

crisi economica latente, ce n'è una sociale che ci può spaventare. Richiamo l'attenzione del Governo su due problemi molto gravi

non usiamo l'autorevolezza del presidente Draghi per far modificare l'atteggiamento della Commissione europea che ci sta penalizzando in maniera grave. È l'ultima occasione per modernizzare il Paese. Siamo assolutamente convinti che questi interventi, nella visione organica dei decreti sostegni e sostegni *bis,* daranno un aiuto alle imprese (specialmente a quelle piccole e medie), alle famiglie e alle fasce più deboli.

Per aiutare le imprese basta considerare il *rating* del merito creditizio pre-Covid. Possibile che non riusciamo a introdurre una norma che obblighi le banche a considerare il *rating* delle imprese prima del Covid e non quello successivo alla pandemia, che sicuramente è peggiorativo?

La Lega ha dato un contributo durante i lavori che si sono svolti in Commissione non soltanto in termini di partecipazione e di determinazione, ma anche e soprattutto di contenuti e dell'importante miglioramento che è stato portato all'interno del provvedimento. Siamo qui per dare

dei lavoratori separati, della TOSAP e degli aiuti ai più deboli e alle imprese. Abbiamo puntato tantissimo su questo e si vede la differenza. Da genovese e da ligure

sulla sponda destra del Polcevera, perché quella è stata una tragedia che tutti noi italiani, noi liguri e noi genovesi, non dimenticheremo mai.

un segno forte e importante per il futuro di quella città, che mai dimenticherà quello che è avvenuto. *(Applausi)*. Credetemi, saranno molti quelli che mai dimenticheranno il modello Genova: a me piace parlare di modello Lega Genova, perché con il Sottosegretario di allora, con il vice ministro Rixi, con Matteo Salvini e con il sindaco Bucci siamo stati in prima linea. Quel modello Genova ancora oggi deve richiamare tutti noi al superamento dei vincoli, dei lacci e dell'impossibilità concreta di fare le grandi opere a causa di questo codice degli appalti che dev'essere riformato, per non dire cancellato e

e siamo per la Gronda e per arginare chi ancora oggi politicamente non vuol fare queste grandi opere. *(Applausi)*. Si passa da lì e lotteremo fino in fondo per la politica del fare e non per una volta a cancellare lo sviluppo del Paese.

leggere la lettera di un medico del 118.

Leggo la lettera di un medico del 118: durante la pandemia solo noi del 118 siamo entrati nelle case delle persone malate di Covid. Eppure, nessuno ci aveva detto come procedere. Ci siamo trovati ad attendere per ore in ambulanza fuori dai pronto soccorso, finché l'ossigeno del mezzo di soccorso non si esauriva. Ci siamo vestiti dalle sei alle otto volte al giorno, imparando come fare guardando i video dello Spallanzani. Ci siamo autotassati per comprare sapone e carta asciugamani. Siamo entrati nelle case di anziani soli, che ci hanno chiesto di preparare i loro indumenti buoni per andare in ospedale. Abbiamo raccolto i loro effetti personali in una borsa, abbiamo etichettato tutto con il loro nome e imparato a trascrivere i numeri di telefono sui referti. Abbiamo chiuso le loro case, prendendo le chiavi. Abbiamo visto migliaia di persone poco prima che morissero. È stato umanamente toccante, bellissimo e terribile al tempo stesso. Eppure per noi non esiste alcun servizio di supporto psicologico. Amo il mio lavoro, ma credo che me ne andrò non appena ne avrò la possibilità, come già hanno fatto molti miei colleghi. È un lavoro pesante, con turni massacranti e livelli di remunerazione inferiori a quelli degli altri medici, che non offre alcuna tutela, come in molti abbiano realizzato nel momento in cui ci siamo ammalati di Covid e non avevamo diritto né all'infortunio, né alla malattia. Il medico che scrive si chiama Roberta Ladisa ed è uno di quegli eroi che hanno permesso al nostro Servizio sanitario nazionale di reggere. *(Applausi)*. Eppure il 118, che è il baluardo della nostra assistenza territoriale, è stato dimenticato in tutti i decreti che abbiamo approvato in quest'Aula. Al 118 non sono dedicati fondi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi però, per la prima volta, in un decreto-legge si parla di 118 e io il decreto-legge sostegni lo chiamo decreto riscatto per il 118. Questi medici, oltre a essere stati dimenticati, in quest'anno hanno anche subito l'ingiustizia di veder richiesta la restituzione dell'indennità per lavoratori a rischio che hanno percepito negli ultimi quindici anni. A questi medici convenzionati è stato decurtato lo stipendio del 25 per 800 euro al mese, perché, in virtù della scarsa chiarezza che regola il loro contratto di lavoro, la Corte dei conti ha chiesto un approfondimento alla regione Campania sull'indennità

in autotutela hanno inviato a questi medici una lettera che chiede la restituzione dell'indennità che hanno finora percepito. Immaginate cosa significa per un medico impegnato nella gestione di questa emergenza ricevere una lettera che chiede di restituire in unica soluzione cifre che vanno dai 70.000 ai 100.000 euro L'effetto chiaramente è stato l'abbandono delle postazioni 118 da parte di molti medici. Pertanto, le ASL campane hanno dovuto fare bandi per assumere medici tramite cooperative, attraverso contratti di lavoro come volontari, e sappiamo che poi questi operatori vengono retribuiti con finti rimborsi di pochi euro. euro. Il rischio era quindi di smantellare un servizio di emergenza che invece è fondamentale per il nostro Servizio sanitario nazionale. Da un anno un anno segnaliamo e denunciamo in tutte le sedi istituzionali questa ingiustizia. Abbiamo depositato qui in Senato due interrogazioni, la prima a febbraio 2020 e la seconda a febbraio 2021, chiedendo al Ministro della salute di porre fine questo scempio e di sollecitare l'aggiornamento dell'accordo collettivo nazionale. Alla Camera il nostro Gruppo parlamentare ha discusso in Aula un'interpellanza e in Regione Campania la nostra vice presidente Valeria Ciarambino si batte al fianco al fianco di questi operatori sanitari da un anno, attraverso atti depositati in Commissione sanità e chiedendo anche il passaggio a contratti stabili per questi medici che sono precari storici. il decreto-legge in esame prevede il riscatto di questi medici, perché, grazie a un nostro emendamento approvato in Commissione bilancio, non dovrà più essere restituita l'indennità finora percepita Confido che questo emendamento sia inserito nel testo definitivo del decreto-legge e sia accolto con favore da tutte le forze politiche, perché le battaglie per i diritti devono essere di tutti. Altre battaglie e sfide dobbiamo combattere assieme per riscattare tutti i nostri eroi, tutto il nostro personale sanitario che - lo voglio ricordare - quest'anno è candidato al premio Nobel per la pace (mi riferisco al personale sanitario italiano). Tra gli eroi da riscattare ci sono, ad esempio, i dottorandi, ai quali purtroppo non siamo riusciti a garantire il raggiungimento del minimale contributivo INPS; ci sono gli operatori sociosanitari, che, dopo aver lavorato nella gestione di tutte e tre le fasi pandemiche, continuano a ricevere lettere di licenziamento. Ci sono i medici di comunità e cure primarie, specialisti che si sono formati per la gestione delle cure primarie e della medicina di comunità e per operare nell'ambito della medicina generale. Eppure, nonostante due decreti interministeriali prevedano che come ambito di azione per questi medici ci sia la medicina generale, questo ancora non è permesso. Avevamo provato a sanare questo *vulnus* con due emendamenti, che purtroppo hanno avuto parere contrario, nonostante la carenza dei medici di medicina generale in questo Paese e la necessità di strutturare le case di comunità, che sono proprio i luoghi in cui questi specialisti dovranno operare. invito, colleghi, è allora davvero quello di unirci per portare avanti battaglie che vadano nella direzione di valorizzare tutto il nostro personale sanitario alla riforma della formazione medica e a quella dell'emergenza-urgenza territoriale), perché tutelare i nostri operatori sanitari significa tutelare il diritto alla salute dei cittadini italiani. A tutti gli operatori sanitari vanno la mia

i nostri relatori per l'ottimo lavoro svolto, sia il collega Manca, sia la collega Toffanin. Il provvedimento che ci apprestiamo a discutere e a votare è il frutto del lavoro di settimane, con cui abbiamo cercato di dare ascolto alle richieste di aiuto che ci provengono ormai da tutte le categorie. Come rappresentanti delle istituzioni, siamo chiamati a a fare tutto il necessario per fornire supporto e sostegno a tutte le categorie colpite, a fronte di una crisi che veramente ha colpito tutti indistintamente. Possiamo e dobbiamo ancora fare molto, ma credo che fino a questo momento abbiamo compiuto un buon lavoro, prima con i decreti rilancio e ristori e ora con il decreto sostegni, al quale a breve seguirà un decreto sostegni Questi provvedimenti sono la chiara dimostrazione del fatto che la crisi non è passata. Siamo ancora in emergenza pandemica e stiamo cercando di rialzarci, anche con l'importante lavoro fatto nel campo delle vaccinazioni, vaccinazioni, per poter dare un po' di sollievo alle attività economiche che sono in sofferenza da troppo tempo, ma anche per poter tornare finalmente a respirare un po' di normalità. Abbiamo lavorato in questa direzione e gli importanti emendamenti approvati ne sono una chiara dimostrazione: l'esenzione integrale del canone RAI per il 2021; ma anche la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga, previsti dalla legge di bilancio la possibilità di anticipare la decorrenza della fruizione dei trattamenti previsti dal decreto sostegni, al fine appunto di consentire la continuità con i precedenti periodi. Vi è poi la concessione di un contributo a favore dei concessionari di aree demaniali marittime, per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento attivo e passivo, che hanno la necessità più più che mai di essere rilanciate. Queste sono solo alcune misure contenute nel decreto che ci apprestiamo a votare, misure che, come Italia Viva-PSI, abbiamo fortemente voluto e su cui abbiamo canalizzato il nostro impegno nel lavoro di queste settimane in Commissione (ne approfitto per ringraziare tutti i colleghi e le colleghe delle Commissioni competenti). Come Capogruppo in Commissione istruzione e cultura, però, penso anche alle misure che riguardano il settore della cultura e dello sport, forse tra le categorie maggiormente colpite dalle restrizioni adottate per contenere il virus. In questo importante lavoro, Italia Viva-PSI ha giocato un ruolo centrale e decisivo. Pensiamo infatti che far ripartire la cultura e il mondo dell'intrattenimento significhi in parte far ripartire la vita e la normalità. È stato approvato il nostro emendamento a favore degli operatori dello spettacolo (qui ringrazio come primo firmatario Riccardo Nencini): si tratta di agevolazioni per le spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività culturali, anche se si sono utilizzati sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, come rappresentazioni teatrali, concerti e balletti. Abbiamo messo in campo fondi utilizzabili come credito di imposta pari al 90 per cento quale contributo straordinario: è senza dubbio una misura importante, soprattutto perché si tratta di un contributo che è compatibile anche qualora le imprese abbiano beneficiato di altri finanziamenti, a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Poi lo sport, che non è stato lasciato indietro, ma era ed è davvero in ginocchio; è un tema su cui ci siamo sempre battuti come Italia Viva-PSI. È stato infatti approvato un altro importante emendamento, che porta la mia prima firma, con cui viene ulteriormente rifinanziato un fondo previsto dal decreto-legge ristori, con uno stanziamento di 50 milioni di euro, per il periodo 2020-2021, per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche. passo in avanti e vigileremo affinché il decreto attuativo della norma preveda che tali risorse siano effettivamente destinate ad associazioni e società che non hanno potuto accedere al contributo a fondo perduto in quanto non titolari di partita IVA. Nello stesso senso va anche la misura, sempre voluta dal nostro Gruppo, che consente il rimborso per gli abbonamenti relativi all'accesso a impianti sportivi di ogni tipo. Come sappiamo, le misure di contenimento adottate in questi mesi per fronteggiare il virus hanno toccato l'intero tessuto economico, ma probabilmente il settore degli impianti sportivi è stato uno dei quelli più colpiti duramente, se non altro perché le chiusure si sono protratte e continuano purtroppo ancora a protrarsi. Peraltro, l'emendamento approvato consente che il rimborso consista, in alternativa alla restituzione del corrispettivo, nell'emissione di un *voucher* pari valore, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale. Si tratta di interventi di grande aiuto per il mondo sportivo, che si trova in affanno per la lunga sospensione delle attività a causa del virus. Il settore dello sport è trasversale e anche noi, come Gruppo, ci siamo mossi per cercare di ascoltare le istanze provenienti da tutti gli operatori che si muovono all'interno di questo mondo. A titolo esemplificativo, è stato approvato un emendamento a favore dei maestri di sci, con il risultato di uno stanziamento di 40 milioni in favore della categoria. È fondamentale sostenere questo settore, così come lo è sostenere il comparto della cultura e dello spettacolo. Ci abbiamo lavorato con passione e impegno; abbiamo lavorato tutti insieme: anche questo è un salto di qualità e una pagina nuova del nuovo Governo e di questo Parlamento. Insomma, credo che siamo consapevoli delle conseguenze disastrose che ha determinato questa epidemia. Ci attende uno sforzo ancora più grande, e il provvedimento di oggi va nella direzione giusta.

per i cittadini che si devono approcciare alla ripartenza. C'è bisogno, insomma, di fiducia e anche di sicurezza, di certezza e di programmazione, accanto a una campagna vaccinale che sicuramente ha fatto un salto di qualità.

dovremmo fare una riflessione ulteriore, maggioranza e minoranza assieme, sperando chiaramente che il monitoraggio ci dia dati sempre migliori e che soprattutto la campagna di vaccinazione possa accelerare

cercando di capire la ragione per la quale siamo arrivati all'ennesimo decreto indennizzi, sostegni o ristori: cambiamo il nome, ma non deve cambiare purtroppo la sostanza. Infatti, prima di giudicare e di commentare, siamo abituati a valutare le ragioni

credo di poter definire Merkel-Macron, perché ormai purtroppo c'è un pensiero unico in Europa: se lo dice la Merkel e lo dice Macron, allora è verità. allora è verità. Peccato però, cari colleghi, che innanzitutto non abbiamo le disponibilità finanziarie di Macron, tantomeno quelle della Merkel. Non siamo coloro che hanno potuto dare indennizzi del 60-70 per cento a quelle partite IVA che avete fatto e state facendo soffrire. Noi siamo quelli - non dimentichiamolo - che hanno dato complessivamente alle partite IVA e alle aziende poco meno del 6 per cento delle perdite. Non dimentichiamolo mai: non il 60 o il 70, ma poco meno del 6 per cento, con

rappresentano di fatto il 3 per cento. Questi sono i numeri veri. Ecco perché la verità Merkel-Macron non si può tradurre in verità in Italia e comunque in verità assoluta. Basterebbe guardarsi intorno, avere il coraggio e l'umiltà di riconoscere i propri errori, signori del Governo; riconoscere i propri errori e non essere cocciuti, insistere, come state insistendo, in questa logica. Penso anche al coprifuoco:

Guardiamo ad altri Paesi, come la Russia, che ha evitato il *lockdown* di autunno e non è messa peggio di noi, tutt'altro. Ma guardiamo più vicino: Stoccolma, una città metropolitana ed europea, che addirittura non ha fatto *lockdown*, ha tuttavia dati molto migliori dei nostri. Guardiamo Madrid - questa è politica - dove vi è stata la vittoria dei popolari anti *lockdown* sulla sinistra socialista spagnola al Governo, che con il *lockdown* voleva rovinare anche Madrid. I popolari hanno avuto il coraggio di dire di no e Madrid ha risposto con un'economia più fiorente e con una sanità migliore della nostra.

e non vi pagherà: se ammetteste i vostri sbagli, qualche volta, sarebbe un bene per voi *in primis* e per il Paese, ricordiamolo.

a un'attiva politica fiscale di massa. Abbiamo tre strumenti da utilizzare: il ravvedimento operoso, l'adesione e la conciliazione giudiziale. Avremmo potuto dire ai cittadini: «Regolarizzate le vostre posizioni fiscali, pagate il 100 per cento delle imposte e vi abboniamo le sanzioni e vi raddoppiamo la rateizzazione da 48 mesi a 8 anni». stata una politica educativa, utile a tutti i cittadini e a tutte le imprese, non come la buffonata dell'articolo 4; avrebbe permesso ai cittadini di mettersi in regola con il fisco, nel tempo giusto e senza essere gravati da sanzioni. dico che siamo un'opposizione costruttiva e perché abbiamo l'onore di poter dire che vi portiamo su un piatto d'argento proposte che potreste fare vostre e che invece, per il fatto che provengono dall'opposizione, vi guardate bene anche solo dal considerare. Altre le risposte che avete dato sui cui contenuti non ci avete ascoltato. Non si potevano utilizzare i 5 miliardi del *cashback* o il denaro impiegato nella lotteria degli scontrini per indennizzare

Non si poteva magari evitare, con la proroga continua degli sfratti, di addossare ai piccoli proprietari il ruolo di *welfare* che spetta allo Stato? Perché oggi il cittadino, che magari ha un paio di appartamenti sui quali vive, comprati con la propria liquidazione o i propri risparmi,

Stato? Voglio pensare poi anche alle risposte che non avete dato in questo decreto-legge e che continuate a non dare. Continuate a far brindare le mafie, cari colleghi.

quindi le critiche che potremmo muovere a questo decreto. Naturalmente le risposte di Fratelli d'Italia, come ho detto, sono tante. Alcune le ho citate. Ricordo anche il tema della liquidità:

e quindi utilizzare la leva finanziaria che permette chiaramente di moltiplicare per sei, sette e otto le garanzie, dando liquidità alle imprese. Questo si doveva fare:

Concludo, però, con una nota positiva e un ringraziamento a quei colleghi trasversali della politica, dal Partito Democratico alla Lega, che hanno voluto supportare una battaglia che stiamo conducendo da circa due anni sul differimento termini dei professionisti. Riconosciamo alle Commissioni riunite di averci approvato un emendamento importantissimo per i professionisti italiani, che finalmente - per ora per la materia Covid, ma ma sono certo che, assieme a voi, arriveremo ad approvare nelle prossime settimane il disegno di legge che è da oltre un anno in lavorazione in Commissione - hanno il diritto di hanno il diritto di potersi ammalare senza dover pagare le sanzioni. Avranno quindi il diritto di essere parificati agli altri lavoratori e agli altri cittadini.

accettare le proposte e le idee dell'opposizione, ne guadagniamo tutti, ma soprattutto il Paese. Non è utile giocare sporco; non è utile volersi arrogare solamente i meriti; bisogna condividerli,

Abbiamo trovato copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a questioni che erano rimaste fuori. Pensate al supplemento di copertura finanziaria concernente tutta la debolezza di categorie del lavoro che abbiamo riconosciuto come invisibili, ancorché fondamentali: i lavoratori stagionali, quelli che hanno prestazioni con ritorno ciclico all'interno delle attività riguardanti la collettività e la moltitudine, come la cultura e lo spettacolo. Abbiamo trovato copertura ai costi fissi delle imprese. È immaginabile una società che ricominci a girare con vigore e fiducia, se non consentiamo alle imprese di superare quegli impedimenti necessitati e imposti dall'ordinamento? Il *lockdown* ha per ragioni riferite al contagio da bloccare. È chiaro che questo ha portato a nudo i costi fissi delle imprese. Abbiamo fatto un lavoro di discernimento laico e lucido nel merito per avere il consenso di tutti. Abbiamo lavorato per fare in modo che realtà tipo l'economia bianca della montagna non riguardasse soltanto i grandi numeri della montagna del Nord, ha una forza di trazione per la collocazione turistica nazionale e internazionale. Attraverso l'attività emendativa di merito abbiamo fatto in modo che si ricomprendesse anche anche la montagna dei piccoli numeri dell'Appennino, che però consente l'offerta turistica del sistema Paese Italia. Abbiamo fatto in modo che anche figure riguardanti l'innovazione della cultura e della ricerca, come i dottori di ricerca, venissero a trovarsi davanti all'opportunità di allungare la propria *expertise* di applicazione nella ricerca e nell'innovazione. Dobbiamo sapere che senza queste risorse dell'innovazione per l'innovazione non ci sarai economia capace di competere sul piano internazionale.

modo abbiamo trovato la maniera per permettere ai Comuni il rispetto della produzione dei documenti contabili per tempo e adeguatamente, perché anche loro hanno patito la guerra la guerra dell'interruzione della normalità e dell'attività dei dipendenti preposti alla cura dei documenti contabili. Lo potranno fare i Comuni entro il 30 settembre di quest'anno, grazie ad un emendamento, che mi ha visto impegnato in prima fila, perché ho visto la fatica di alcuni Comuni, rinnovati di recente, che non ce la facevano. E non è possibile che la regola della pubblica amministrazione prevalga rispetto alla vita reale. *(Applausi)*. A questo proposito voglio mettere in evidenza un dato: abbiamo anche fatto sì che le norme sanzionatorie dell'Unione europea, riguardanti la vita delle imprese, a proposito di una norma lucidissima, che volle Gino Giugni al tempo del migliore periodo degli anni Novanta, quando cioè si passò dalla formazione del dire a quella del fare, per cui i giovani venivano introdotti nel circuito del lavoro attraverso i contratti di formazione e lavoro.

Abbiamo presentato un emendamento e lo abbiamo istruito favorevolmente, con la lucidità della politica, perché la regola, il diritto pubblico e la decisione pubblica non possono uccidere la vita reale e così si è consentita la rateizzazione.

A quei 150 miliardi di euro adesso si aggiungono i 248 miliardi di euro del *recovery plan* e le risorse del prossimo settennio della programmazione, come Stato membro

Non è possibile che ci vogliano settantadue mesi per mettere a regime la qualità di un progetto. In Italia abbiamo fatto passare un messaggio sbagliato e sbilenco. Sblocca cantieri? No! Prima di tutto serve uno sblocca progetti, in maniera tale che il progetto abbia la comanda dell'opera da farsi. Dobbiamo ricostituire le competenze nella pubblica amministrazione, per fare in modo che ciò che si vuole

da un terreno in possesso, che venne dato loro da Mussolini, ad un terreno che poi sarebbe stato affrancato, secondo le parole pronunciate dai vertici di Palazzo Chigi nel corso di cento anni. Siamo ancora in attività istruttoria, nonostante il Parlamento abbia deliberato e legiferato. Questa è la prova simbolo di come a volte la pubblica amministrazione arrivi a divorare, ad ostruire, ad assumere un atteggiamento da mammalucco, nei confronti di progetti che riguardano la vita reale.

non togliere la salvaguardia del rispetto della trasparenza, del diritto penale e della *par condicio*, ma occorre fare in modo che i pronunciamenti degli enti terzi arrivino per tempo, perché questo tipo di lavoro, finanziato dalla risorsa pubblica, consentirà alle imprese di avere digitalizzazione e cablaggio, nei rapporti tra progetto di vita dell'impresa e sistema della PA e consentirà alle scuole di avere la continuità dell'offerta formativa, come all'università. Pensate anche al bisogno di telemedicina,

ci sarà bisogno di organizzare la continuazione dell'offerta formativa, educativa e della sanità a distanza. Tutto questo richiede investimenti, ma anche attività decisionale nell'immediatezza, misurazione della quantità e della qualità dei risultati e valutazione. Abbiamo conosciuto lo *smart working*, una forma organizzativa imposta per necessità, ma dobbiamo anche riorganizzare i carichi di lavoro per fare in modo che si tratti di lavoro e che non sia la negazione del lavoro. Tutto questo richiede che si continui a legiferare nel merito, come abbiamo provato a fare nell'attività riguardante il primo decreto-legge sostegni: un'attività che ha tolto di mezzo la polemichetta, l'atteggiamento di interesse di parte. Sono molto soddisfatto, per esempio, per il lavoro che siamo riusciti a mettere a segno a proposito dei settori deboli della cosiddetta economia della collettività, della consistenza numerica. Pensate agli impianti di sciovia, agli impianti della montagna: sarebbe immaginabile che si liberino dalla debolezza senza l'aiuto pubblico? C'è un settore - quello delle realtà aeroportuali non ha conosciuto alcun tipo di sostegno. C'è stato un tentativo di aiuto nella legge di bilancio in esercizio quest'anno; ancora, però, deve arrivare a destinazione. Dobbiamo aiutare le società aeroportuali altrimenti perderemo la connettività aerea, che significa velocità per le economie, facilità negli spostamenti. Il quadro delle questioni lo dobbiamo tenere a mente sapendo che non è finita, che il valore di 1.700 miliardi riguardanti il nostro PIL non si ripristina né con i 32 miliardi già deliberati né con i 40 che delibereremo. C'è bisogno di mettere a sistema una condizione di premura e di aiuto che davvero recuperi quello che abbiamo dovuto interrompere. Ce la dobbiamo mettere tutta, dobbiamo fare in modo che la pubblica amministrazione sia un alleato della vita reale e dobbiamo fare in modo che le misure destinate alla formazione e all'innovazione siano davvero a disposizione di tutti i luoghi... *(Il

Signor Presidente, siamo oggi qui riuniti a discutere del decreto-legge sostegni, che elargisce 32 miliardi per il ristoro di tutte le perdite subite dalle aziende in questo periodo di pandemia.

vengono stanziati 150 milioni per il recupero dei *gap* formativi. Purtroppo, però, il piano del ministro Bianchi, che aggiunge a questi 150 milioni altri 320 a sul PON e altri 40 per le povertà educative (per un totale complessivo di 510 milioni di euro),

specialmente delle scuole superiori. È qui che si è accumulato un *gap* formativo che di sicuro non potrà essere colmato con un piano estivo che prevede esclusivamente attività laboratoriali, di supporto, di sostegno psicologico, nonché di orientamento:

incoerenza anticipano anche la chiusura delle scuole, aprendo agli scrutini già dai primi di giugno.

oltretutto non prevede alcun impegno nell'impugnativa di tutte quelle ordinanze illegittime delle Regioni, che hanno previsto la scuola *à la carte*. In pratica, le famiglie possono scegliere se far seguire ai figli i corsi da casa oppure se farli seguire in presenza, in questo modo vanificando anche quest'ultimo mese di scuola che, purtroppo, non andrà a influire minimamente sul miglioramento della formazione dei nostri studenti.

ministro Gelmini a suo tempo, investendo per approfondire la qualità dei piani di studio, per ridare un senso alle discipline che si affrontano nei piani di studio delle scuole di ogni ordine e grado e poi per ridurre il numero degli alunni per classe. A settembre, infatti, se ci troveremo nella stessa condizione, con un numero invariato di studenti per classe nelle stesse strutture deficitarie che noi, purtroppo, abbiamo nel nostro patrimonio immobiliare scolastico, rischieremo di perdere un altro anno di formazione per i nostri studenti. Non esiste alcuna misura di ristoro per tutto questo lavoro perso, per la scuola italiana e per gli studenti; una generazione compromessa in maniera quasi irreversibile, visto che, comunque, non c'è la volontà di porre rimedio a tutto questo. I *gap* formativi non si risolvono con misure *spot* da 150

alla senatrice Toffanin e al senatore Manca, ai Presidenti delle due Commissioni, senatori D'Alfonso e Pesco, e al Governo. Sono state due settimane veramente importanti e di intenso lavoro.

categorie che sono state assolutamente devastate, in questo anno, da questa crisi economica e dall'uragano della pandemia. Noi abbiamo oggi il diritto-dovere di aiutare queste categorie in difficoltà. Abbiamo resistito

500.000 vaccinazioni al giorno. Oggi ci siamo finalmente riusciti. Questa sarà oggi la nostra arma per combattere la pandemia e uscire finalmente dalla crisi. L'impatto economico è stato devastante, soprattutto per il tessuto produttivo del nostro Paese, che si basa su piccole e medie imprese che non hanno un'autonomia

una linea coerente all'opposizione, coerente oggi all'interno del Governo, perché anche in passato abbiamo votato gli scostamenti di bilancio e lo abbiamo fatto nell'unico interesse dei cittadini italiani. Questo è stato sempre il nostro scopo. Ai cittadini italiani oggi - usando una metafora - va data una coperta per ripararsi ancora dalla notte che è ancora fonda e poi va data anche la benzina, anche la benzina, perché in questo momento dobbiamo riaccendere i motori, dobbiamo ripartire, dobbiamo ritornare a correre, a vivere e a volare e finalmente a salutare - speriamo quanto prima

con i dovuti ringraziamenti ai relatori, perché hanno valorizzato il lavoro di tutti i colleghi e dei Gruppi e non era una cosa scontata. Ringrazio i Presidenti, che hanno supervisionato tutta l'analisi del decreto e che invito a voler arginare, per i prossimi decreti,

ma con dei tempi stabiliti, quindi purtroppo anche in questo caso abbiamo dovuto fare una sola lettura. Ma proprio perché è una sola lettura occorre, soprattutto nel momento di sintesi finale, avere il tempo per evitare che possano rimanere delle imperfezioni e dei piccoli errori che poi andranno sistemati in altri provvedimenti. Ringrazio il Governo, in particolare il vice ministro Castelli e i sottosegretari Durigon e Bini. tutti gli uffici che hanno supportato con l'abituale professionalità tutti i lavori della Commissione. Ma veniamo ai contenuti. Effettivamente il lavoro ha visto una convergenza dei vari Gruppi su temi prioritari e quindi c'è stata un'unica azione rispetto all'esenzione COSAP-TOSAP. La Lega con grande forza ha chiesto l'esenzione del canone RAI per quegli esercizi pubblici che sono stati chiusi e tale richiesta è stata condivisa anche dagli altri Gruppi. È stato fatto, a mio avviso, un lavoro molto importante. In molti interventi ho parlato dell'importanza della variabile tempo; c'è stata una sinergia con le Regioni per arrivare a migliorare, sia in termini di tempo che di efficacia, il lavoro. Mi riferisco in particolare a quanto uscito all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni rispetto al riparto per la montagna. C'è stato quindi un lavoro preparatorio importante. Come è stato detto da molti colleghi, con un ordine del giorno chiediamo al Governo che nel decreto-legge venga incrementato di 100 milioni il Fondo per la montagna. Non solo, anche rispetto agli accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria, il fatto che gli adempimenti previsti dal comma 492 potranno decorrere dal 2022, farà in modo di non bloccare il riparto del Fondo sanitario nazionale 2021 e avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Anche questo è un ottimo traguardo.

che le associazioni e le società sportive dovranno onorare nonostante la sospensione della propria attività a causa della pandemia. Tante volte è dato per scontato, ma vorrei ricordare che l'attività che svolgono le associazioni e le società sportive

il proprio stato di salute mentale e fisica, ma coinvolge anche un discorso di socializzazione con un grande effetto sulla capacità di lavorare in squadra e stare insieme. Il blocco di queste attività pertanto una ferita per tantissime persone, soprattutto giovani. Il secondo intervento sullo sport molto importante concerne la possibilità di avere la proroga per l'entrata in vigore dei contratti sportivi. C'è assoluta consapevolezza che le società sportive non siano ancora pronte; la proroga al 31 dicembre 2023, quando la scadenza sarebbe stata il 1° luglio 2022, è stata un'ottima realizzazione. Ci sono anche misure più piccole che la Lega ha voluto portare come proposte emendative che danno un segnale preciso. Sto parlando, ad esempio, della somma

molti problemi li hanno anche gli agenti di polizia penitenziaria, che devono essere attrezzati giustamente per poter affrontare momenti di grande emergenza e di pericolo. Questo è un piccolo segnale, a nostro avviso, molto importante. Non solo, abbiamo anche voluto dare un segnale per quei lavoratori, genitori separati, che a causa della pandemia hanno avuto difficoltà perché hanno perso il lavoro o comunque hanno dovuto tenere chiuse le proprie attività; un Fondo di 10 milioni di euro potrà aiutare loro al pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli fino a 800 euro. Anche questo

in questo anno trascorso, con il problema della raccolta pubblicitaria e della possibilità di sopravvivenza. Questo è quindi un altro segnale molto preciso.

Vorrei fare un ultimo riferimento a un argomento importante, grave, che ha colpito tutti in questi giorni. Dopo i festeggiamenti del 1° maggio, quando forse si è parlato di

Temo che in molti casi le difficoltà economiche abbiano comportato

dovrebbe tutelare tutti i lavoratori, qualunque ruolo essi abbiano. È una battaglia che ancora dovremo combattere tutti insieme.

queste risorse così copiose e nella possibilità di far riprendere tutte le attività, con la giusta prudenza, perché forse molte volte si fraintende. Nessuno dice: liberi tutti, non importa. La prudenza e il senso di responsabilità ci devono essere, ma proprio per prudenza e per senso di responsabilità dobbiamo permettere a tutti i lavoratori, a tutte le famiglie, di riprendere una vita normale, di riprendere il lavoro, che non dà solo sostentamento ma anche dignità, il senso della vita,

per la stesura del secondo decreto-legge sostegni di prossima emanazione. Dal lavoro e dalla lettura degli emendamenti di tutti i Gruppi è emersa la comune volontà di sostenere imprese, lavoratori e famiglie in questo che speriamo sia l'ultimo frangente di pandemia. Questo è ancora il momento di salvare con tutti i mezzi necessari il lavoro e la capacità produttiva del Paese. L'abbiamo fatto finora, nell'anno appena trascorso. L'abbiamo fatto nelle settimane scorse con il lavoro nelle Commissioni e lo ha fatto il Governo sul solco tracciato dal Governo Conte, con un impiego di risorse in un solo anno mai visto prima nel nostro Paese. Quando la pandemia sarà terminata e riprenderemo finalmente a vivere, non dobbiamo però dimenticarci il senso di profonda inquietudine provato quando abbiamo visto le nostre strade strade e piazze vuote; quando abbiamo visto i nostri negozi, i nostri bar e i nostri ristoranti chiusi; quando abbiamo visto le nostre piccole imprese private della possibilità di vivere. Non dobbiamo dimenticarci che la vitalità delle nostre città è data ancora dalle piccole attività economiche. Non dobbiamo dimenticarci quanto è emerso in modo drammatico nell'anno appena trascorso. I nostri piccoli imprenditori e le partite IVA, nonostante da sempre abbiano sostenuto il tessuto economico e anche sociale del Paese, sono ancora la fetta più importante di popolazione priva delle più elementari forme di garanzia che spettano di diritto a ciascun lavoratore. Con l'ultima legge di bilancio abbiamo previsto una nuova forma di cassa integrazione per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (ISCRO), in via sperimentale. Dopo la pandemia dovremo stabilizzare questa misura estendendola a tutte le categorie di lavoratori autonomi. È nostro dovere farlo. È un principio di giustizia sociale. Oggi siamo chiamati a un salvataggio di emergenza con le misure che ci apprestiamo ad approvare. Anche questo è un nostro dovere. tante le ciambelle di salvataggio previste nel testo originario del decreto sostegni e sono tante anche le nuove misure introdotte dal Senato nelle Commissioni finanze e bilancio, di cui hanno parlato i colleghi ieri e oggi in discussione generale, tra cui l'esonero per alberghi, bar e ristoranti dalla prima rata IMU, dal canone RAI, dalla tassa di occupazione del suolo pubblico; l'esonero per i proprietari dal pagamento delle imposte sugli affitti non riscossi; i ristori alle *start-up* - di cui ringrazio il collega, primo firmatario, senatore Dell'Olio - che non hanno ricevuto finora indennizzi. Le misure aggiuntive sono tante e sono tutte straordinariamente rivolte a sostenere imprese e lavoratori in difficoltà. Ci tengo a richiamare, tra i tanti emendamenti approvati, tre che hanno introdotto nuove tutele per i lavoratori dei porti industriali, tra cui il porto canale di Cagliari. all'emendamento a mia prima firma, sostenuto dalla vice ministro Alessandra Todde e dai colleghi parlamentari sardi del MoVimento 5 Stelle, tra cui la collega Evangelista, e agli emendamenti dei senatori Emilio Floris di Forza Italia e del senatore Giuseppe Luigi Cucca di Italia Viva; colleghi che ringrazio, come sardo, per aver espresso anche in questa occasione la comune volontà di operare, al netto delle diverse sensibilità politiche, per il bene della nostra Isola. ancora l'emendamento del MoVimento 5 Stelle a prima firma del collega senatore Mario Turco, che ha esteso la cessione anche ai crediti di imposta del Piano nazionale transizione 4.0, una delle misure più finanziate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Grazie a questa novità, abbiamo di fatto introdotto una sorta di superbonus imprese, consentendo alle imprese di cedere liberamente i crediti d'imposta per investimenti in innovazione e formazione e in ricerca e sviluppo e, quindi, non solo di usarli in compensazione, come era previsto finora. La novità rende ancora più vicina e a portata di mano una tra le principali proposte economiche del MoVimento 5 Stelle, ovvero il potenziamento di una piattaforma elettronica per certificare e far circolare i crediti di imposta immessi nel sistema. A questo proposito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva che stiamo portando avanti nelle Commissioni finanze di Camera e Senato, è emerso il suggerimento di autorevoli auditi di slegare dalla dichiarazione dei redditi il tema della redistribuzione del reddito e dell'incentivo agli investimenti e agli acquisti per le spese cosiddette meritorie. Secondo questi esperti, è piuttosto discutibile utilizzare il sistema delle detrazioni e deduzioni in dichiarazione redditi, perché impoverisce la base imponibile Irpef, tagliando spesso fuori dai benefici i cosiddetti incapienti. Sarebbe invece più efficiente un sistema di sussidi diretti nel caso di interventi redistributivi, commisurati - ad esempio - alla dichiarazione ISEE. In questo senso, occorre una riflessione sull'impiego di crediti d'imposta cedibili quali sussidi diretti; crediti d'imposta slegati dal sistema delle detrazioni e deduzioni che sappiamo tanto danno hanno fatto al nostro sistema fiscale. I crediti d'imposta cedibili possono essere una valida soluzione di sussidi e sostegni diretti, per diverse ragioni: funzionano; garantiscono un'erogazione immediata ai beneficiari; comporteranno un esborso da parte dello Stato, ovvero un minor gettito, soltanto una volta ottenuti gli effetti positivi anche per il gettito dello Stato. L'utilizzo dei criteri d'imposta potrebbe essere una soluzione a saldo zero per le casse dello Stato, ma con effetti dirompenti per l'economia, per l'ambiente e per le famiglie (vedi il superbonus). il mio intervento con l'argomento con cui ho iniziato. Il nostro è un Paese di microimprese. Non facciamoci sedurre da modelli che non ci appartengono. È un modello che sicuramente mostra elementi di debolezza, di forte debolezza - ad esempio - nei confronti dei colossi *web*, ma è anche un sistema che ha sempre dimostrato una capacità di reazione e resilienza superiore a sistemi di altri Paesi. Le nostre piccole imprese sono sempre state in grado di innovarsi e adattarsi alle mutazioni del mercato. L'indipendenza, la capacità di resilienza e la fantasia delle nostre microimprese sono lo specchio del nostro modo di essere. Anche il nostro superbonus è una misura italiana, un'intuizione italiana, perché coniuga rilancio e sviluppo della vera economia verde, efficientamento energetico, miglioramento del nostro patrimonio edilizio e anche dell'umore degli italiani, perché parliamo del bene più prezioso che hanno: la casa. Gli emendamenti al decreto-legge sostegni, che hanno esteso la cedibilità anche ad altri crediti d'imposta, sono un segno importante. Occorre prima o poi mettere in ordine il sistema dei crediti cedibili anche attraverso lo sviluppo della piattaforma realizzata recentemente dall'Agenzia delle entrate per certificare questi crediti, rendendoli quindi certi e sicuri per lo Stato e spendibili per l'acquisto di beni e servizi. Questa potrebbe essere una strada tutta italiana di autofinanziamento: tutta italiana esattamente come le nostre piccole imprese. *(Applausi)*.

con il loro contributo, portare alla nostra attenzione e a quella del Governo ancora proposte ed evidenziare delle criticità che possono comunque essere costruttive in vista dei futuri provvedimenti, a cominciare dal decreto-legge sostegni-*bis.* È vero: quello che stiamo per approvare è un buon provvedimento; non è un provvedimento di certo risolutivo, vista la pandemia ancora in corso; considerate le risorse limitate che abbiamo avuto a disposizione rispetto allo scostamento votato lo scorso gennaio,

Questo Governo non può di certo accontentare tutte le richieste e soddisfare le esigenze e le gravi criticità che emergono nel nostro Paese. È vero: sono stati presentati 2.852 emendamenti al provvedimento, ma ciò non significa che la maggioranza abbia bocciato il decreto-legge in esame. Anzi, credo sia stata, invece, data la possibilità

dai cittadini, attraverso i loro rappresentanti e tutte le associazioni che sono stati auditi nelle Commissioni finanze e bilancio. Poi, però, la responsabilità di questa maggioranza si è esplicitata nel lavoro di grande sintesi che è stato portato avanti, prediligendo misure di ampia portata, che hanno trovato una grande convergenza e hanno evitato che le ulteriori risorse a disposizione del Parlamento finissero disperse in tanti rivoli, ovviamente impercettibili e inefficaci a livello di intervento. Certo, si poteva fare meglio. Si può fare di più - come ho già detto nella mia relazione - e noi siamo pronti a impegnarci anche per il futuro. È tuttavia vero che questo Governo non è la continuazione del Conte II: mi pare evidente che abbia dimostrato una grande discontinuità, anche per il fatto che il PNRR, sul quale poggia il futuro nostro e di tutto il Paese, sicuramente è stato migliorato ed è stato presentato nei termini previsti. L'Europa aveva bocciato il precedente, ma il Governo Draghi è riuscito a presentare un progetto che può rimettere rimettere in moto tutto il sistema Paese. È anche vero che, con il Governo Draghi, il Parlamento - come abbiamo dimostrato con questo provvedimento - ha lanciato un segnale importante, perché ha riacquistato il proprio ruolo nel processo legislativo, dando un forte contributo e soprattutto riuscendo ad incidere sul provvedimento

usa più la logica del *bonus*, che vogliamo dimenticare, ma si parla di incidere sui costi fissi delle imprese sono state chiuse e non hanno potuto usufruire dei servizi sui quali noi vogliamo portare delle agevolazioni.

a chi riceve il contributo. È per questo che abbiamo impegnato il Governo a intervenire con la moratoria dei mutui, ma anche creando nuovi fondi di garanzia dello Stato, perché l'impresa per ripartire ha bisogno di liquidità. Noi Noi abbiamo anche chiesto al Governo di poter procedere con le riaperture, che devono essere effettuate al più presto, perché solo con il lavoro si potrà far ripartire il nostro sistema.

bisogno di implementare il piano delle vaccinazioni. Abbiamo bisogno di riaprire le nostre attività e di immettere liquidità per fare investimenti. Queste saranno le ricette che ci daranno la garanzia di poter di poter rimettere in moto l'economia e il nostro sistema. Credo che con il decreto in esame abbiamo dato un bel segnale, perché ci siamo innestati in tale logica. che finalmente porteremo a casa un risultato con questo che sarà il primo di tanti provvedimenti. E vorrà essere anche una denotazione del Governo Draghi, che finalmente ha ascoltato il Parlamento, ponendosi in una logica diversa per cercare di dare risposte in una situazione veramente drammatica e preoccupante, e insieme, con lo stesso spirito di collaborazione che ha visto unita questa maggioranza, potremo cominciare a dare qualche segnale di ripartenza.

penso che la discussione generale abbia consentito a noi tutti di trovare ambiti di riflessione che vanno molto al di là del decreto in conversione. Come avevamo detto nelle relazioni di presentazione del provvedimento, il nostro lavoro si è concentrato non solo a definire le misure utili per la conversione, ma anche e soprattutto a a indicare al Governo gli indirizzi fondamentali per la definizione del nuovo decreto sostegni-*bis*. Tuttavia, colleghi, parto da un primo dato che vorrei chiarire almeno tra di noi: non credo credo sia utile al Paese introdurre la polemica sul coprifuoco. Questo decreto ha destinato oltre 5 miliardi al Sistema sanitario del nostro Paese; oltre 2,8 miliardi per l'acquisizione dei vaccini e sappiamo tutti qui dentro - non c'è nessuno che non lo sa - che la velocizzazione delle vaccinazioni rappresenta la prima misura economica per uscire dalle limitazioni individuali ed economiche che ovviamente la pandemia ha imposto al nostro Paese. Non c'è nessuno che non vuole superare dunque il coprifuoco. Dobbiamo però tener conto che dobbiamo lavorare con grande attenzione per aprire le attività in sicurezza, perché il nostro obiettivo è aprire, e non richiudere tra pochi mesi. Il nostro obiettivo è liberare il Paese in sicurezza

di aprire polemiche assurde per dare l'idea che ci sia una contrapposizione tra chi vuole liberare il Paese dalle limitazioni e chi, invece, vuole costringere il Paese nelle limitazioni. È un dibattito assurdo e inspiegabile perché, se velocizzeremo il piano di vaccinazione come stiamo facendo, raggiungendo 500.000 vaccinazioni giornaliere - sono diverse dalle 100.000 che facevamo pochi settimane o pochi mesi fa - riusciremo ad arrivare, acquisendo i vaccini, (ci sono 2,8 miliardi destinati) a un'immunità di gregge che ci metterà nelle condizioni di uscire in sicurezza dalle limitazioni. L'ambizione di questo Paese deve essere però più grande, colleghi. Credo che sia molto importante sottolineare qui che sono state individuate alcune risorse anche per portare l'Italia all'interno delle produzioni vaccinali. Il nostro Paese deve avere l'obiettivo di proteggere i cittadini da future varianti e anche da future pandemie. E, per fare questo, abbiamo bisogno - come abbiamo indicato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - del primo e più importante investimento sulla dimensione territoriale del sistema sociale e sanitario. Abbiamo visto, infatti, quanto sia difficile curare le persone all'interno di fenomeni pandemici e non possiamo non tener conto di questa situazione. L'esperienza pandemica ci porta a ritenere l'investimento nella dimensione territoriale la primaria operazione da fare per mettere in sicurezza l'Italia. Altro che polemiche da coprifuoco! Lavoriamo insieme da subito per progettare un nuovo sistema sociale e territoriale che si prenda cura e torni a restituire centralità alla medicina di base e territoriale, che è uscita dal *radar* dell'alta specializzazione dei grandi ospedali e dei grandi luoghi di ricerca. Non voglio mettere in contrapposizione la ricerca dei grandi ospedali, ma abbiamo visto che, senza una medicina territoriale più forte; senza una medicina telematica che porti a casa delle persone le cure necessarie; senza una medicina di base nuovamente centrale, non riusciremo a proteggere il Paese da future varianti pandemiche. Lo dico perché trovo sbagliato, anche da parte di Fratelli d'Italia, continuare a insistere su questa polemica perdendo di vista l'obiettivo cruciale che il Paese deve avere, e cioè garantire una sicurezza fondamentale alle famiglie e alle imprese anche di fronte al probabile arrivo di nuove ondate di nuove varianti e anche di nuove pandemie. Questa deve essere la sfida di un grande che ha uno dei sistemi sanitari universali più forti in Europa e nel mondo. Credo che dobbiamo partire da questo ragionamento perché da qui si capisce il giusto investimento che abbiamo fatto sull'architrave del nostro Paese. Le piccole e medie imprese sono l'architrave del nostro Paese. Chiunque legge l'economia italiana sa che la piccola e media impresa è l'asse portante della nostra economia. Era doveroso un intervento sui costi fissi. Abbiamo introdotto elementi di novità rispetto al passato: abbiamo superato i codici Ateco; tutti insieme e senza litigi politici risorse fondamentali per aiutare le piccole e medie imprese. Sono centinaia di migliaia le attività che giustamente oggi hanno uno Stato più vicino. Abbiamo tolto di mezzo incrostazioni e attriti che potevano anche generare conflitti sociali e mettere in difficoltà il sistema dell'ordine pubblico e della sicurezza del Paese. Aver destinato oltre 430 milioni di euro alla riduzione dei costi fissi è stata una scelta politica giusta che non ha colore e rappresenta la maggioranza che sostiene questo Governo. Ha determinato anche l'indirizzo per ulteriori risorse sulla liquidità delle imprese

territoriale. La crisi pandemica ha aperto nuovi squilibri e ampliato la forbice tra chi non ce la fa e chi ce la fa. Abbiamo un tema di fragilità sociale nella dimensione territoriale molto ampio, al quale si connettono tutte le questioni alle quali abbiamo cercato di dare alle quali abbiamo cercato di dare una prima risposta, compreso il tema difficile gli sfratti. Non è una sconfitta: è un primo tentativo per dare una risposta, che però non può non avere al suo fianco anche la dimensione sociale della portata della sfida. infatti, chi lo sfratto lo subisce dentro dinamiche di povertà acquisite all'interno della fase pandemica e c'è chi lo sfratto lo ha acquisito perché già prima non voleva pagare il canone e, quindi, ci sono dinamiche sociali molto delicate anche all'interno degli sfratti. Abbiamo cercato

al settore turistico e alle imprese turistiche. Abbiamo sempre detto, sin dal primo giorno, che è una delle filiere che ha bisogno di un'attenzione particolare perché rappresenta un ambito di potenziale crescita del prodotto interno lordo del nostro Paese. L'Italia è una piattaforma naturale sul piano culturale e ambientale. Per le sue bellezze architettoniche e la qualità della vita non ha rivali nel mondo. Dunque è evidente che dobbiamo cominciare a ragionare per filiere: non siamo tutti uguali, non tutte le dinamiche economiche si scaricano in maniera proporzionale.

Dunque dobbiamo mettere in campo investimenti e favorire gli investimenti privati. Se vogliamo che questo settore resti italiano - come è giusto che sia - abbiamo bisogno di spazi ulteriori, di crediti di imposta e di meccanismi fiscali favorevoli al rilancio degli investimenti.

A queste dinamiche dobbiamo unire l'investimento fatto sul lavoro, le riforme necessarie per riorganizzare gli ammortizzatori sociali e la necessità di spostare risorse dall'assistenza alle politiche attive, dobbiamo essere sempre consapevoli che un reddito di formazione diventerà decisivo, nei prossimi anni, per accompagnare una nuova crescita, e lo si farà attraverso un'importante riforma degli ammortizzatori sociali. gli elementi decisivi dell'universalità del Sistema pubblico sanitario, con la forza sociale ed economica che contraddistingue il nostro Paese. Credo che, in questa dinamica, con l'immunità di gregge, con l'uscita dalla pandemia, nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con le riforme, l'Italia abbia tutte le condizioni per uscire dalla crisi.

inquadrare l'argomento e di evidenziare le iniziative di Fratelli d'Italia, per migliorare un decreto-legge, che sicuramente non ci vede particolarmente entusiasti.

un entusiasmo forse esagerato per aver scritto, su un ordine del giorno, i *desiderata* per il prossimo decreto-legge.

un entusiasmo forse un po' eccessivo, che non solo stride con il fatto che la maggioranza abbia presentato 2.500 emendamenti, a dimostrazione che il provvedimento non piaceva particolarmente a nessuno e non solo alla minoranza di Fratelli d'Italia, che ne aveva presentati Ciò stride soprattutto con lo sconforto e lo scoramento che c'è fuori da questo palazzo, dove tante categorie produttive pagano, pagano, come tutti i cittadini - e non solo - le limitazioni anticostituzionali della libertà, come l'assurdo coprifuoco, che continua a persistere nonostante non ci sia alcuna evidenza scientifica del fatto che il virus morda di più dopo le 22, rispetto a prima. E non solo questo: pagano quelle attività produttive che fino ad oggi hanno tirato la carretta di questa Nazione; pagano sulla propria pelle anche le chiusure e le limitazioni della propria attività. Cito due esempi: gli agriturismi, che erano oggetto di emendamenti *bipartisan*, sono gli unici che non ricevono nemmeno un indennizzo, perché non si è scorporata la loro attività di agriturismo da quella agricola. Questo credo sia emblematico di come sia prestata poca attenzione soprattutto a quelle categorie che riempiono le nostre mense e le nostre cucine di prodotti sani, tipici, e costituiscono l'ossatura di quel *made in Italy* di cui tutti ci riempiamo la bocca, ma che ben pochi, poi, cercano di supportare in maniera concreta.

- al di là delle questioni e delle diatribe interne al Governo tra chi ha una visione più privatistica della soluzione del problema e chi, come il Governo precedente e la Regione Veneto, magari intravedeva una prospettiva di strategicità

come sono sicuro che lei, Ministro, vuole scongiurare - non siano i tanti lavoratori e soprattutto le tante famiglie che intorno all'Acc ed Embraco in Piemonte vivono e lavorano. Credo che il giudizio che possiamo dare, anche dopo il dibattito che abbiamo ascoltato in Aula, sia assolutamente insufficiente, come lo sono state le misure; insufficiente come sono i giudizi che arrivano da tante categorie. Noi siamo sempre stati a disposizione. Ringrazio i relatori, sia la collega Toffanin che il collega Manca, per la disponibilità e le aperture che hanno avuto nei confronti dell'opposizione, consci -come siamo - di avere sempre lavorato non per far crescere nelle percentuali il nostro partito - anche se è oggettivamente un dato di fatto anche quello - ma soprattutto con il solo interesse, di far crescere questa Nazione che noi - contrariamente magari a qualcuno di voi - non vogliamo certo vedere né soffrire né tantomeno asservita alle logiche europee di Francia e Germania.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

dalle Commissioni riunite, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

La seduta è ripresa. Alla luce dell'intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento, salvo nelle parti che riproducono gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite che la Presidenza si accinge a dichiarare improponibili e alle condizioni di seguito indicate. Gli emendamenti 11.7 (testo 2) e 21.0.2 sono improponibili. è proponibile a condizione che venga riformulato in senso aggiuntivo all'articolo 35 del decreto-legge. L'emendamento 39.30 (testo 3) è proponibile limitatamente ai capoversi 1-*bis* e 1-*quater* e a condizione che l'applicazione dello stesso sia circoscritta nel tempo e cioè fino al limite massimo del 31 dicembre 2022. L'emendamento 39.0.56 è proponibile in una nuova riformulazione e condizione che l'applicazione dello stesso sia circoscritta nel tempo, cioè fino al limite del 31 dicembre 2022. L'emendamento 39.0.66 (testo 2) è proponibile a condizione che l'applicazione dello stesso sia circoscritta nel tempo e cioè fino al limite del 31 dicembre 2022.

successivamente. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge

presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente che è fin d'ora autorizzata a convocarsi. Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia. Avverto che

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge sostegni. La seduta riprenderà alle ore 15,30 o comunque al termine della seduta della Commissione bilancio chiamata ad esaminare i profili finanziari dell'emendamento. Per la discussione sulla fiducia sono stati assegnati cinque minuti per ciascun Gruppo. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato altresì il calendario dei lavori della prossima settimana. La giornata di martedì 11 sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento alla Commissione affari costituzionali chiamata ad esaminare il decreto-legge sul contenimento dell'epidemia Covid-19, vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici. La discussione di quest'ultimo provvedimento avrà inizio nella seduta di mercoledì 12, con inizio alle ore 10. Il calendario dei lavori prevede, inoltre, nella giornata di giovedì 13

Per la discussione delle mozioni sono previsti per ciascun Gruppo cinque minuti nella discussione e dieci minuti per le dichiarazioni di voto, oltre ai cinque minuti attribuiti per l'illustrazione delle mozioni. Eventuali mozioni abbinate dovranno pervenire entro le ore 18 di martedì 11 maggio. Sempre nella giornata di giovedì 13 maggio, alle ore 15, si svolgerà il *question* *time* con la presenza dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e del turismo. Mercoledì 12, alle ore 9, è convocata la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati per procedere alla sua costituzione.

di accelerare i tempi. Per quanto riguarda questa Presidenza, le 16,15 è l'orario limite entro cui si può far aspettare l'Aula

consenso quasi bulgaro, eccetto la mia parte di emiciclo, ancora, a distanza di tempo, si arrovella su un emendamento e non trova la quadra. A pagarlo siamo noi che siamo bloccati in Aula da oltre un'ora, con continui rimandi. Credo sia bene stigmatizzare questo comportamento che certo non fa bene al Parlamento.

Ho informato il Presidente del Senato del ripetersi della richiesta di ulteriori rinvii; le ho chiesto di farmi sapere in proposito

Presidente, credo che a questo punto una regola di buona amministrazione della gestione dell'Assemblea dovrebbe essere quella di dire che non è serio arrivare con modifiche di emendamenti che non riusciremo a capire; né riusciremo a capire in quali parti il testo che andiamo a votare viene rimaneggiato. Per questa ragione, signor Presidente, le rappresento la necessità di rappresentare al Governo che forse è preferibile rinviare tutto a martedì, perché si voti consapevoli di quello che votiamo.

sia più serio che il Parlamento sia informato e sappia quello che vota. Come noto, non faccio più parte della maggioranza, essendo stato cacciato insieme ad altri colleghi il 17 febbraio, per non aver votato la fiducia al presidente Draghi. Non parlo quindi come esponente della maggioranza, essendo relegato nel Gruppo Misto.

è stata espunta dal Ragioniere generale dello Stato. Ma chi era il precedente Ragioniere dello Stato? Era il ministro Daniele Franco. Allora bisogna

Presidente, abbiamo sempre una parola sola. Non siamo certo noi quelli che tradiscono gli accordi, quindi ribadisco la nostra disponibilità a iniziare, nonostante non ci sia il testo, stigmatizzando però quanto avvenuto, ossia un ritardo di un'ora e mezza dovuto solo ed esclusivamente a diatribe interne alla maggioranza, che ci hanno visto addirittura abbandonare la Commissione, visto il comportamento assolutamente inusuale e che certo lede fortemente le nostre prerogative parlamentari.

lo abbiamo dimostrato con il superbonus edilizio al

che ciò che è stato fatto in Commissione non lo possiamo accettare. Il MoVimento 5 Stelle non ritrae la mano in questo momento alle persone che aspettano il decreto sostegni; ma da domani

dimostra la presenza di una maggioranza che sta sfiorando, ogni momento di più, il ridicolo.

che addirittura il Capogruppo del primo partito che sta in questo Parlamento non conosca le regole parlamentari e non sappia che sto facendo un intervento

il senatore De Bertoldi - lo dico a chi non l'ha capito - non sta intervenendo sull'ordine dei lavori. *(Commenti)*. Stia buona, stia zitta, Il senatore De Bertoldi sta intervenendo sulla questione di fiducia e sta svolgendo un intervento politico in cui può esprimere le sue opinioni.

Santangelo, lei è espulso dall'Aula. Sospendo la seduta per cinque minuti.

questa volta sulla questione di fiducia, se lo desidera - il senatore Licheri, che potrà esprimere tutte le opinioni che ritiene nell'occasione e nel modo previsti

mattina con un auspicio di trasversalità e collaborazione, che era tanto atteso e importante in un momento così difficile per il Paese e nell'interesse di tutti gli italiani, al di là delle fazioni, dei partiti e delle ideologie politiche.

Orbene, poiché, come il collega De Carlo ha detto prima, siamo abituati ad avere una parola sola, ci aspettavamo che, con la stessa serietà con la quale abbiamo chiesto alla maggioranza la fiducia su tre emendamenti,

voleva garantire la flessibilità e che, in un momento di grande difficoltà per i nostri territori, le Regioni non fossero rigidamente costrette a impiegare i fondi per spese con voci precise e dettagliate, ma che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome potessero utilizzare quel denaro che i vari decreti emergenziali avevano dato per le necessità che si appalesavano sul momento. Faccio anche un esempio, perché i cittadini devono capire, citando il caso di quando sono state destinate risorse, dai decreti emergenziali, per l'assunzione di personale sanitario.

abbiamo dunque chiesto di fare in modo che quel denaro, che non si è potuto spendere rigidamente per l'assunzione, potesse ad esempio essere speso per utilizzare quel personale sanitario in modo temporaneo.

che ha cercato di rispondere alle esigenze delle Regioni italiane, che sono anche quelle del popolo italiano, offrendo risposte ai cittadini in modo immediato e non vincolato, ci dovesse essere coerenza.

che potrebbe consentire alle nostre aziende di rilanciarsi e di rilanciare il nostro tessuto economico. Adesso dobbiamo cominciare a guardare oltre i sostegni e i sussidi: dobbiamo assolutamente farlo, ma dobbiamo guardare al futuro. Abbiamo constatato che, tra la serata di ieri e la mattinata di oggi, l'emendamento che concerneva la cedibilità dei crediti d'imposta delle imprese per la vendita dei beni strumentali nell'ambito del piano Transizione 4.0 ha

inizieremo un tavolo, perché quell'emendamento inizi il suo percorso che lo porti al decreto-legge sostegni-*bis*. Interloquiremo e abbiamo avuto garanzie importanti da parte del Governo perché il tema non venga accantonato;

abbia sparato a due pescherecci italiani, ferendo uno dei comandanti. Questo episodio è particolarmente grave, perché ricordiamo tutti che, pochi mesi fa,

Che il fatto si sia ripetuto - addirittura, sembra che ci siano feriti a bordo - è a mio avviso particolarmente grave, perché ci chiediamo tutti dove sia la Marina italiana.

Stiamo affrontando l'approvazione di un decreto-legge che è più di una manovra di bilancio. C'è una grande urgenza; in 5a Commissione abbiamo fatto approfondimenti doverosi,

sono priorità per tutti i Gruppi politici. Su questo abbiamo interloquito tutti con il sottosegretario Durigon, quale ha garantito che l'interlocuzione continuerà, proprio perché questi tre temi possano essere affrontati nel decreto-legge sostegni due o comunque possano trovare una formalizzazione

sono emendamenti che impattano in maniera incredibilmente importante sulla vita delle aziende, delle cooperative e dei lavoratori. Rimane una priorità e penso che oggi ci siamo presi tutti l'impegno di concentrarci, perché venga trovata una soluzione.

che le imprese avrebbero potuto convertire in denaro, dopo aver acquistato beni strumentali per l'innovazione tecnologica, ma sono stati tolti anche tutti quegli strumenti che, parimenti a questo, consentivano la cedibilità dei crediti. È stata tolta la cedibilità dei crediti per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici, che era invece stata approvata con un emendamento a prima firma Mininno, sottoscritto da tutti i rappresentanti di L'Alternativa C'è, e anche

tutti coloro che non sono stati toccati dalla crisi e a carico soprattutto di coloro che invece hanno aumentato i loro profitti con il Covid-19, ovvero i colossi del *web* e tutti coloro che hanno ottenuto enormi guadagni da questa crisi, gestendo le piattaforme informatiche per gli acquisti *on line*. line*. È stato tolto tutto questo, ma invece c'è il condono. Ci sono i regali, incrementando i fondi per le emittenti locali, e gli acquisti per le divise antisommossa. Alla luce di questo, chiedo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: vi siete resi conto con chi vi siete messi a governare? Avete capito che questo Governo

che si è reso disponibile ad aprire un'interlocuzione per risolvere le questioni tecniche che esistono e che la Ragioneria ha sollevato. Cerchiamo quindi di tenere insieme tutto. Questo è lo spirito del Governo che stiamo sostenendo e mi preme che non si ripetano le condizioni in cui abbiamo lavorato nell'ultima ora in Commissione bilancio.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, preso atto: della rassicurazione del Governo secondo cui la circoscrizione della portata temporale degli emendamenti 39.30 (testo 3), 39.0.56 (testo 39.0.66 (testo 2), richiesta come condizione di proponibilità di tali proposte emendative, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica; con specifico riferimento all'emendamento 39.30 (testo 3), capoverso 1-*quater*, l'attuale formulazione, che ne delimita l'applicazione temporale al 31 dicembre 2021, appare comunque conforme alla condizione di proponibilità; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: siano soppressi l'articolo 1-*ter*, l'articolo 1-*quater*, il comma 3-*bis* dell'articolo 24, il comma 11-*octies* dell'articolo 30 e l'articolo 40-*ter*; l'articolo 1-*sexies* sia così riformulato: "l. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall'articolo 1, comma 493 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica "Covid 19", all'articolo l, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "La citata Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità", sono sostituite dalle seguenti: "La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a 14 unità, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Resta fermo il limite di spesa, per l'anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018."; all'articolo 12-*bis*, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021"; all'articolo 18-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "di concerto" siano inserite le seguenti: "con il Ministero dell'economia e delle finanze all'articolo 19-*bis*, al comma 1, siano soppresse le seguenti parole: ", come rifinanziato dall'articolo 41"; - all'articolo 26, comma 1, le parole: "le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea", ovunque ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: "le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"; all'articolo 30-*septies*, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190";

si provvede quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e quanto a 1,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

Signor Presidente, è davvero importante lo sforzo compiuto con il provvedimento in esame, che segna soprattutto un salto di qualità nell'individuare le categorie e i criteri di erogazione delle risorse. Innanzitutto - ed è giusto ricordarlo - si archiviano i codici Ateco per introdurre il principio delle perdite di fatturato. È un passo in avanti, anche se il periodo di riferimento non tiene in adeguata considerazione quelle imprese che nel primo trimestre del 2021 non hanno incassato un solo euro. Comprendo la preoccupazione sulle lungaggini burocratiche, ma c'è una vasta platea che percepirà aiuti non corrispondenti alle effettive perdite. Questo rammarico è compensato dall'annuncio del ministro Franco, che su nostra proposta si è impegnato a introdurre presto un nuovo periodo di riferimento per indennizzare adeguatamente le aziende che hanno subito gravi perdite anche con il nuovo anno. Ed è in parte compensato anche dal buon lavoro svolto in Commissione, che ha introdotto migliorie e ha arricchito il testo; per questo ringrazio i presidenti di Commissione Pesco e Alfonso e ringrazio i rappresentanti del Governo, *in primis* il vice ministro Castelli, e lo *staff* di MEF e di Ragioneria dello Stato. l'ennesima conferma del valore del lavoro parlamentare e del modo in cui, attraverso il confronto, si possono costruire provvedimenti più vicini alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Penso alle misure sui costi fissi, dalla prima rata IMU alla cancellazione della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, agli interventi sul canone RAI e sull'Irpef per i canoni di locazione non percepiti. Penso alle norme sui liberi professionisti, tra cui la sospensione delle sanzioni per i mancati adempimenti legati alle malattie, ma anche alla proroga IRAP, alle tutele sui mutui e sull'assegno di mantenimento al consolidamento delle risorse per il turismo termale, ai contributi a fondo perduto per i bus turistici. Si può continuare ancora con i 40 milioni per i maestri di sci, con le importanti risorse per gli impianti di risalita, con i 230 milioni per gli operatori economici di montagna nel capitolo complessivo del riordino degli interventi sulla filiera della neve. Si tratta davvero di tante misure e di un massiccio intervento, che vede anche l'accoglimento di una serie di nostre proposte per i tirocini e il potenziamento delle attività extrascolastiche nei nostri territori, la correzione del buco normativo sulla CIGO e la proroga della CIG, le semplificazioni burocratiche per l'accesso agli esoneri contributivi da parte delle aziende e delle imprese agricole. È importante ricordare anche le altre misure, che non sono state oggetto di particolari modifiche, ma che costituiscono i pilastri del provvedimento: dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali al pacchetto di aiuti per le partite IVA, alle risorse per gli albergatori e i luoghi della cultura, per i lavoratori termali, per lo sport dilettantistico, per l'agricoltura, per i Vigili del fuoco, nonché il fondo importantissimo per garantire il funzionamento degli enti locali. Presidente, questi miliardi rappresentano un'ulteriore tappa per garantire la tenuta sociale e per accompagnare il nostro sistema produttivo nel dopo pandemia. Conosciamo tutti la gravità della situazione e sappiamo che questo non sarà l'ultimo intervento, che presto sarà necessario un altro scostamento di bilancio e che siamo dentro un percorso che rinnova continuamente le sue sfide. In tal senso, è molto importante l'ordine del giorno di maggioranza che introduce già le questioni che dovranno essere affrontate nella conversazione del decreto 100 milioni di ulteriori risorse per sostenere la filiera della montagna, un massiccio intervento a favore dei lavoratori stagionali che non godono più di alcuna forma di ammortizzazione sociale, l'accesso al credito, garanzie moratorie prorogate a fine anno per le imprese, il credito di imposta sul canone di locazione, l'esenzione degli oneri contributivi per la cultura e lo spettacolo, la riduzione della Tari per le imprese. Mi auguro che tutto questo rientri nella cornice di una revisione dei periodi di cui dicevo prima, ma spero anche che si avvii una riflessione su quella che sarà la nostra economia una volta usciti dalla pandemia. Questi quattordici mesi hanno scosso le fondamenta del nostro sistema economico, portando alla luce limiti e ritardi, ma in molti casi anche una grande capacità di resistenza e di adattamento alla nuova fase. Sarebbe però un errore ritenere la pandemia come una parentesi. Siamo in un salto d'epoca, che apre a sfide inedite, come ha ben compreso l'Unione europea con le missioni legate al piano, e che richiederà anche un salto nel pensare il mondo del lavoro e il sistema produttivo. Uscire dalla pandemia - cito il presidente Draghi - non sarà come riaccendere la luce; alcune attività economiche dovranno cambiare, anche radicalmente. Per questo bisognerà lavorare sul binomio flessibilità-sicurezza sociale, rendendo, da un lato, più dinamico il mercato del lavoro e, dall'altro, rafforzando gli ammortizzatori sociali. Dovremo cioè immaginare un campo più agile dentro un perimetro dove continua a farsi sentire la presenza dello Stato. Dovremo cioè definire con sempre maggiore chiarezza il modello di Paese verso cui vogliamo tendere partendo, e non finendo, dai progetti del *recovery fund*. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento. membri del Governo, colleghi, in verità non riesco ad esprimere giubilo, come alcuni interventi che ho ascoltato su questo provvedimento, se non a condizione che da ora in poi noi tutti qui si lavori per la crescita. Oggi, grazie al Governo Draghi e alla campagna vaccinale del generale Figliuolo, ci sono le condizioni per lavorare finalmente sulla crescita economica e sullo sviluppo, per sviluppare domanda, investimenti pubblici e investimenti privati, ed è esattamente quello che dovrebbe occupare il Parlamento.

un presupposto non sufficiente; è un presupposto semplicemente necessario. È stato quindi sicuramente necessario aiutare le imprese in difficoltà con la cassa integrazione per i dipendenti, con la CIG, ed estendere questi provvedimenti anche alle *start-up*, come abbiamo fatto in fase di conversione. Così come importante è stato aiutare i settori più colpiti, come il turismo e la ristorazione, cercando di abrogare imposte, tasse, canoni, come abbiamo fatto con il canone RAI, con la prima rata dell'IMU e con l'occupazione degli spazi pubblici. Una misura, quest'ultima, importante nel momento in cui i ristoranti possono partire, possono ricominciare a lavorare per cui devono beneficiare di questa misura. Importante è anche l'intervento sulla montagna. Ho vissuto vari anni in montagna e so che perdere tutta la stagione invernale vuol dire perdere il 90 del fatturato. Per gli alberghi, per gli impiantisti, per i maestri di sci in questo e nel prossimo provvedimento ci sarà molta attenzione. Abbiamo lavorato sui settori finora esclusi

al *tax credit* sulla cultura, un settore straordinario che in questa misura ha il seme per poter ripartire. E penso poi alle televisioni locali, che hanno fatto informazione di prossimità, tenendo compagnia alle persone chiuse in casa e rassicurandole.

Quindi sì, ritengo sicuramente che questo sia stato un provvedimento importante, ma non condivido le celebrazioni per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché questi due tasselli, il decreto-legge sostegni e si collocano in un quadro macroeconomico che resta comunque molto fragile, tutto da ridisegnare e da trasformare secondo quanto abbiamo scritto nel PNRR, ma che è da portare a terra. secondo luogo, perché 32 miliardi più 40 miliardi sono un indebitamento netto importante e noi non possiamo essere soddisfatti nel dire che che volentieri redistribuiamo risorse a debito. Questo è un messaggio culturale che personalmente non condivido, un messaggio di politica economica che dovrebbe essere esattamente il contrario: noi economicamente dovremmo dire che le risorse le generiamo e poi le redistribuiamo. Questa è una condizione data, in cui la politica espansiva è semplicemente obbligata, ma non possiamo compiacercene e nemmeno abituarci. abbiamo molto presente ciò che abbiamo votato nel DEF quindici giorni fa. Il DEF ci ha detto tre cose molto importanti sull'indebitamento netto, sul rapporto debito-PIL e sul PIL.

Sul rapporto debito-PIL al 159,8 per cento, ci ha detto che, sì, ci sarà un percorso di rientro e che in dieci anni torneremo al livello enorme di rapporto debito-PIL che avevamo prima del Covid-19. Ciò vuol dire che anche tra dieci anni l'Italia non avrà gli strumenti per far fronte a una sicuramente non auspicata, ma comunque da prevedere dal punto di vista economico, nuova crisi.

Noi sappiamo che ci sarà un rimbalzo nel 2021 del 4,5 o del 4,8 per cento, ma che già dal 2023 torneremo ad avere un tasso di crescita inferiore al 2 per cento. Io dico che questo tasso di crescita è troppo basso, anche se lo consideriamo è troppo basso per immaginare di ridurre il debito con questo strumento e per dire che il PNRR farà davvero la differenza solo perché ci sono 248 miliardi

ho ascoltato l'altro giorno le parole del ministro Colao, il quale ha detto che i fondi del PNRR sono una condizione, ma non sono certo una garanzia di successo. Ha dato un messaggio a tutti noi in quest'Aula (e quello che è successo solo un paio d'ore fa è particolarmente emblematico): ci ha detto che la vera sfida è la trasformazione dell'Italia; la vera sfida sono le risorse, altrimenti l'Italia non ce la fa. Per fare tutto questo serve coesione in quest'Assemblea, serve lavorare assieme, per dare benzina all'unica cosa che fa davvero la differenza, che sono le conoscenze e le competenze, per usare quel mezzo che può portare a terra il PNRR che è la pubblica amministrazione. Anche la pubblica amministrazione deve affrontare una sfida per essere *partner*: meno controlli formali *ex ante*, più controlli *ex post*. Bisogna lasciare andare avanti le iniziative, gli investimenti. Pertanto, per votare a su questo provvedimento di mera spesa, dopo un anno di provvedimenti in *deficit*, e per non sentirsi particolarmente superficiali, dobbiamo dobbiamo garantirci l'un l'altro in quest'Aula che, d'ora in poi, lavoreremo per riformare, per trasformare, per creare valore, cioè ricchezza, per creare posti di lavoro. *(Applausi)*. Da questo punto di vista Italia Viva-PSI può garantire il suo massimo impegno, da partito riformista quale è. Ci sono momenti, signor Presidente, in cui vale la pena pensare e agire contro corrente. Come diceva sant'Agostino, giusto è giusto anche se nessuno lo sta facendo, e sbagliato (come accontentarsi di spendere a debito) è sbagliato anche se lo stanno facendo tutti.

dell'insufficienza di questo decreto-legge, che non ci convince per nessun motivo, come opposizione non abbiamo voluto intralciare il percorso parlamentare a suon di ostruzionismo, ma, da opposizione responsabile quale siamo, sia nella Commissione bilancio che in quella finanze, che hanno lavorato a questo provvedimento, abbiamo dato la massima disponibilità nel tentare di contribuire a migliorare il testo. Siamo soddisfatti che questa nostra correttezza istituzionale ci sia stata riconosciuta in modo *bipartisan* da tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento.

Questo Parlamento sta diventando talmente irrilevante che addirittura, qualche minuto fa, a conclusione della discussione sul voto di fiducia, si pensava di poter mettere in voto questo provvedimento senza che fosse ancora arrivato il testo alla Presidenza del Senato.

hanno esordito dicendo che c'è una netta discontinuità rispetto al passato. Perché dico questo nel metodo? Noi ci eravamo illusi che si potesse arrivare ad un provvedimento, come il Governo aveva anticipato, con tre letture parlamentari

Questa è la conferma che la democrazia parlamentare per questo Governo, come per il precedente, è diventata un *optional* piuttosto che un dettato costituzionale. Per quanto riguarda il merito, il decreto sostegni, come i vari decreti ristori 1, 2, 3, 4, e 5, non sostiene e non ristora assolutamente nulla, a dispetto del suo nome, e non fa che rinviare la ripresa economica del Paese a sempre futuri decreti in attesa di approvazione. Abbiamo detto fin da subito che questo decreto non bastava alle imprese, stremate da tredici mesi di epidemia e da tante restrizioni. Ma come si può pensare, Presidente, di risarcire un'azienda dandole, nella migliore delle ipotesi, il 5 per cento delle perdite che ha subito in un intero anno?

Altrimenti, con la modalità con cui si sta andando avanti, non solo servirà un decreto sostegni-*bis*, che come sappiamo la settimana prossima verrà approvato dal Consiglio dei ministri, ma serviranno tanti altri decreti e scostamenti che il Parlamento dovrà dovrà fare. E queste vostre restrizioni sono diventate ormai anacronistiche e persino più severe dell'anno appena passato. In pratica, come dicono i proverbi, si stava meglio quando si pensava di stare peggio, perché almeno lo scorso anno - se ce lo ricordiamo - al termine del *lockdown*, che è stato il 18 maggio 2020 (quindi sarebbe tra un paio di settimane), non c'era il coprifuoco, non c'erano le restrizioni folli dei ristoranti aperti solo negli spazi esterni; non c'era la pretesa di continuare a tenere piscine e palestre chiuse ad oltranza. E sapete cosa è successo alla fine del *lockdown* prima dell'estate? Nulla. Si andava incontro all'estate, i casi di contagio si erano mantenuti bassi, nonostante non ci fossero le misure restrittive che abbiamo avuto oggi e che tutti conosciamo. Allora ci domandiamo: perché, quando abbiamo una campagna vaccinale in corso così imponente, che tra l'altro sta andando bene in questi ultimi giorni (e di questo chiaramente siamo molto felici), felici), continuate a imporre queste misure che non sono restrittive, ma addirittura punitive? Quindi, noi di Fratelli d'Italia ribadiamo la nostra linea. Non c'è miglior sostegno che consentire le riaperture; certamente, riaperture fatte in sicurezza e con con protocolli anche rigidi, ma riaperture che non sono più rinviabili. Il Governo si deve assumere la responsabilità di compiere questo atto, perché vede, Presidente, se non si fa questo, qualcuno si dovrà pur assumere la responsabilità delle chiusure per le attività che, giorno dopo giorno, stanno morendo. E noi riteniamo che non si possa continuare a rinviare. In questi giorni nelle Commissioni - come dicevo prima - ci avete detto di tutto e di più, che tutto ciò che non entrava in questo decreto - è ormai una litania che sentiamo da più di un anno - sarebbe entrato nel prossimo. Sempre questo si dice

Non si può affidare al Piano nazionale la cura di tutti i mali della Nazione. Certo, il Piano nazionale è un'opportunità che non ci sarà più; è una sfida con la storia; è un appuntamento al quale il nostro Paese deve farsi trovare pronto e questo è il punto. Servono, però, le riforme, altrimenti non ci sarà ripresa; non ci saranno finanziamenti e non ci saranno investimenti. Senza le riforme non ci saranno i risultati che sono stati indicati nel Piano.

Siccome di queste riforme ancora non si conoscono neppure le linee guida, temiamo che il vero Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà ancora tutto da riscrivere. Passando ai lavori che abbiamo fatto in Commissione con riferimento Grazie in caso di malattia Covid per i professionisti. Per la prima volta nella storia nazionale non solo i dipendenti, ma anche i professionisti avranno la possibilità di potersi ammalare senza avere grandi problemi. Penso anche all'emendamento che prolunga i lavori per la messa in sicurezza del territorio, per il dissesto idrogeologico dei Comuni e, in particolare, dei piccoli Comuni. Grazie a un nostro emendamento c'è stato il differimento di termine che ha consentito ai Comuni di poter recuperare i milioni di euro che il Governo aveva concesso loro con provvedimenti. L'emendamento sugli operatori della montagna dei colleghi La Pietra e De Carlo consentirà una più equa ripartizione delle risorse stanziate tra le diverse località sciistiche. Sono tutte risposte a temi di forte attualità.

Signor Presidente, autorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, esame è il primo vero provvedimento che emana questo Governo. Si tratta di un provvedimento importante. Abbiamo apprezzato il metodo, l'approccio corretto, il confronto serio e concreto nell'interesse del Paese. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai relatori che tanto si sono impegnati per individuare utili soluzioni per il nostro Paese. Manca, alla senatrice Toffanin, ma anche ai presidenti Pesco e D'Alfonso, che hanno gestito bene i lavori su questo provvedimento delicato. È un ponte ideale È un ponte ideale perché lo scostamento di bilancio fu votato con il precedente Governo. Individuammo con il ministro Gualtieri i fondi necessari perché c'eravamo ovviamente resi conto della drammaticità della situazione del nostro Paese. Avevamo l'esigenza di trovare nuove risorse. All'epoca era molto difficile. Lo abbiamo fatto tutti insieme e l'Assemblea in quell'occasione ebbe modo di dare dimostrazione di responsabilità, che non sempre ho visto, anche in questo dibattito. Era gennaio lo scostamento di bilancio. Dopo c'è stata la crisi di Governo. Abbiamo perso tempo e bisogna chiedere scusa agli italiani. Gli italiani hanno difficoltà a comprendere la lentezza dei meccanismi della politica: c'è stata una crisi, si sono persi due mesi e ora bisogna recuperare. Il contributo però è reale e positivo e il Senato ha dato - a mio avviso - un grande apporto, accurato e intelligente, con la disponibilità messa dal Governo nelle nostre mani.

Il Parlamento ha avuto modo di ascoltare gli italiani e le loro difficoltà, quelli che soffrono e hanno vissuto e stanno vivendo la crisi sulla loro pelle, quelli che rischiano il posto di lavoro lavoro e devono combattere quotidianamente per difendere la loro impresa. E lo abbiamo fatto con grande attenzione, ottenendo risultati importanti. Penso - ad esempio della prima rata dell'IMU, alla sospensione della tassa di occupazione del suolo pubblico fino a fine anno, o all'esenzione dell'Irpef sui canoni di locazione non percepiti ed è molto importante anche la proroga dell'IRAP al 30 novembre. esame non sarà un provvedimento esaustivo e sufficiente per accompagnarci fuori dalla crisi. Abbiamo messo a disposizione le risorse per fronteggiare la vicenda difficilissima e ancora oggi complicata del virus e della pandemia e tutto quello che era necessario per procedere all'acquisto e una campagna di vaccinazione efficiente ed efficace, che ormai si avvia a dare risultati importanti e concreti. concreti. Signora Presidente, per noi esiste una sola politica che porta all'interesse del nostro Paese, composta da più azioni

attenta, deve procedere speditamente, ma avere attenzione alla salute pubblica, perché non ci possiamo permettere dei ripensamenti o dei provvedimenti che andrebbero a inficiare tutti gli sforzi fatti fino ad oggi. sono poi gli aiuti e il supporto per le imprese, per gli italiani, per i cittadini, per i lavoratori e per tutti coloro che sono in difficoltà, fino ad arrivare alle riforme strutturali, che il Parlamento dovrà presto attuare.

ma sappiamo che non sarà sufficiente e il Governo è già pronto. Credo che nei prossimi giorni, al più tardi la prossima settimana, ci sarà il nuovo provvedimento da 40 miliardi di euro. Non è solo questione

e distribuire ricchezza. Abbiamo quindi chiesto e ottenuto, come Partito Democratico e con tutte le forze di maggioranza, un ragionamento ampio consistente, che guarda avanti. E lo abbiamo fatto con gli strumenti parlamentari che sono a disposizione e, dunque, con gli impegni precisi che il Governo ha preso con noi, col Parlamento e quindi con l'Italia intera. Voglio rammentare il credito di imposta per le locazioni commerciali, l'esonero della Tari, le maggiori risorse ai Comuni e alle famiglie in difficoltà economiche. il disagio psicologico dei minori, che è un tema rilevante, che abbiamo posto e che abbiamo intenzione di portare avanti e di far adeguatamente sostenere anche in termini economici. Non dimentichiamo gli investimenti,

2; il tempo è diventato ormai una variabile rilevante per il futuro del nostro Paese. Siamo costretti a chiedere al nostro Governo di fare presto, di fare bene e di fare tutto quanto sarà necessario per permetterci di cogliere e raccogliere la sfida del futuro. In questo quadro generale, con il decreto-legge sostegni 2 arriveremo a rendere operativo - anche grazie agli anticipi che il presidente Draghi ha ottenuto - il *recovery plan*. La discussione è stata approfondita, attenta. Abbiamo dovuto mettere tutto il peso dell'autorevolezza del nostro Governo e del Presidente del Consiglio affinché si potesse procedere il più velocemente possibile. salvo qualche episodio - inclusi quelli odierni - ha dato dimostrazione e capacità di confronto. Ho apprezzato il contributo che è arrivato

che abbiamo dimostrato nell'attività emendativa durante queste giornate difficili possa essere d'esempio. Ci vuole responsabilità, ci vuole

semplicemente non ci possiamo permettere di utilizzare provvedimenti così importanti come questo per il nostro Paese per guardare ai sondaggi e fare scelte tattiche. *(Applausi)*. Dobbiamo pensare solo al futuro dell'Italia. Signora Presidente, in conclusione, gestione dell'emergenza sanitaria e soprattutto vaccinazioni da fare bene e velocemente; riaperture progressive in sicurezza per essere pronti alla stagione estiva, senza timore; apertura al turismo internazionale, come Draghi ha dimostrato di volere fortemente; difesa delle imprese, tutte le imprese, con tutti gli strumenti possibili; supporto agli investimenti privati e pubblici, anche con incentivi; varo immediato del partenza del *recovery plan*; trasformazione ecologica e digitale. Ecco ciò per cui stiamo lavorando: un'Italia che riparta, più verde, più moderna, più giusta, che non tema il futuro sul fronte economico, su quello sociale e - perché no? - anche su quello dei diritti, cari colleghi. La stagione dell'amore per la nostra comunità nazionale non muore mai. Il PD conferma il voto favorevole e la fiducia al nostro Governo.

vorrei partire da una buona notizia: l'amministrazione Biden ha preso una posizione fondamentale relativa alla

Su questo ci siamo battuti. Il Senato ha espresso pareri importanti in siffatta direzione. Sono molto soddisfatto che oggi Draghi abbia assunto una posizione in questa direzione. Dobbiamo chiedere all'Europa di prendere la stessa posizione alla prossima riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio. Insieme a tutti i Gruppi - ringrazio anch'io i Presidenti delle Commissioni e i relatori - abbiamo fatto un lavoro non semplice,

la questione della montagna, la TOSAP e la COSAP, la questione del canone RAI, la questione dei professionisti, la questione relativa ai canoni non percepiti a favore di quei proprietari che, in questo modo, non dovranno, giustamente, pagare le tasse:

che - intendiamoci - forse mai come in questa occasione tutti i Gruppi, anche l'opposizione di Fratelli d'Italia, sulle questioni fondamentali

che ci sono ancora sul lavoro stagionale (agricoltura, turismo, spettacolo) e per quello che attiene i lavori discontinui, i lavori ciclici, i lavoratori cosiddetti invisibili.

non sarei stato convinto - per esempio - nel non mettere al centro il credito d'imposta per gli affitti commerciali a fronte delle categorie che stanno pagando di più di tutte le altre il prezzo della crisi e del *lockdown*. Lo abbiamo fatto.

non erano lo strumento giusto e che bisognava andare non sul mese, ma sull'anno. Vi sono ancora alcune questioni che io pongo. decreto sostegni 2 deve affrontare tre problemi, oltre a quelli che il Governo ha già detto che della perequazione. Esiste un problema di perequazione tra imprese e soggetti: alcuni hanno preso di più e altri hanno preso di meno. Peraltro, quelli che hanno preso di meno non di rado sono quelle imprese che hanno pagato il prezzo più alto: commercio, ristorazione, turismo,

nell'impossibilità oggi - è una cosa assurda - di usare la cassa integrazione, perché sono di derivazione dell'appalto di un'altra impresa. Questi buchi vanno risolti. Poi, c'è il tema di come governiamo la questione dei licenziamenti. Noi avevamo chiesto di prorogare

Usiamo le parole del presidente Draghi: è un condono ed è un errore gravissimo per il messaggio che diamo agli italiani,

fare un lavoro di spalmatura del debito e dare più tempo alle imprese per affrontare la questione. Noi

Ci deve essere una verifica attenta sulla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Va riformata la riscossione

Diversamente, il rapporto di cittadinanza tra gli italiani e questa Repubblica sarà sempre in crisi e diventerà un problema democratico. Attenzione: abbiamo fatto un buon lavoro, ma c'è ancora tanto e tanto da fare. Avremo modo di confrontarci sulle riforme su cui si gioca la svolta di questo Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, chiediamo al Governo un *triplete* stile Mourinho, visto che è tornato di moda. Il *triplete* non può essere calcistico, ma deve essere basato sul successo con i vaccini (che stiamo registrando) e con i quattrini (che stiamo auspicando). fa il presidente Draghi ha detto che in tempi del genere i soldi si danno, non si prendono. Il terzo obiettivo è quello delle aperture: gli orari, le palestre, il *wedding* - potremmo chiamarlo matrimonio, invece che in altro modo - le piscine e tante altre attività che attendono risposte, senza dimenticare il travaglio della ristorazione, del commercio e di altri. Abbiamo avuto più Figliuolo, meno altre persone. Perfino un romano, Bertolaso, ha reso più rapidi i milanesi nei vaccini. *(Applausi)*. In genere accadeva il contrario, mentre è stato un romano a velocizzare una Regione che ammiriamo tutti per la sua nota efficienza.

ha lavorato molto per ribadire la centralità del Parlamento. La centralità del Parlamento c'è anche nelle difficoltà che nel pomeriggio ci sono state, la centralità è anche la fatica di quel che c'è, di quel che ci sarà e di quel che ci sarebbe dovuto essere. essere. Vediamo così che sulla TOSAP, sulla COSAP, sul blocco dell'IMU ci sono state decisioni importanti e consentite anche a noi del Gruppo Forza Italia di rivendicare

ringrazio il ministro Brunetta che ha annunciato poco fa l'apertura del rinnovo contrattuale per il comparto sicurezza-difesa il 14 maggio. Ancora, abbiamo presentato emendamenti per le società sportive, per la proroga delle deleghe al 31 dicembre

per le attività turistiche danneggiate, l'intervento sugli istituti di case popolari, riguardanti l'IVA e il riconoscimento dell'ecobonus, gli interventi che hanno riguardato l'IMU, le macchine agricole le istituzioni che si occupano dei non vedenti, l'azione per quanto riguarda gli impianti sportivi gli interventi sulle *startup* a fondo perduto, di cui si è occupato insieme ad altri colleghi il senatore Damiani, la montagna, gli sgravi Irpef per i canoni di locazione, gli interventi sul canone RAI delle strutture ricettive, la proroga del versamento IRAP al 30 settembre le vicende degli sfratti. Sugli sfratti, vorrei dire che noi riteniamo positivo quanto è avvenuto, ma si può migliorare l'azione. Non siamo i cattivi che vogliono sfrattare i deboli e non siamo deboli con i cattivi, ci sono sfratti decisi prima dell'emergenza Covid e anche il diritto di proprietà fa parte dei diritti che vanno tutelati *(Applausi)*. Riteniamo, quindi, che il meccanismo introdotto rompa l'immobilismo,

e, quindi, a intervenire sulle partite IVA e noi rivendichiamo la difesa dei professionisti del commercio, delle piccole e medie imprese, del popolo delle partite IVA, che sappiamo hanno sofferto molto più di altri settori, ma con qualche garanzia occupazionale o di salvaguardia sociale maggiore (il turismo, gli alberghi, tutte le che ancora attendono risposte). La vera risposta, però, sono i vaccini e le aperture, in cui noi crediamo, senza demagogia ma con molta determinazione. Quell'ordine del giorno per il prossimo decreto impegna la maggioranza misure per le imprese ad alta intensità di lavoro, ad affrontare i temi di erogazione del credito alle piccole e medie imprese con proroghe, con moratorie ulteriori e poi ancora interventi sulla Tari, che certamente deve essere sospesa per chi non può pagare una tassa su rifiuti che non ha prodotto per la chiusura delle attività. Ci sono i temi dei lavoratori stagionali, delle fiere, dei minori, della cultura,

ad avere tempi più lunghi per il rimborso dei prestiti, tassi ragionevoli e un sostegno vero all'economia reale. Guardiamo quindi molto anche al futuro, alle risorse che serviranno per la sicurezza ed anche per un capitolo che è stato trascurato,

prestiti di lunga durata a basso tasso di interesse aiutino le piccole e medie imprese italiane e che si utilizzi meglio lo scostamento di bilancio. Sono proposte che abbiamo avanzato e che all'interno del Governo e della maggioranza faremo valere anche nei prossimi provvedimenti. Pensiamo ancora alla difesa del 110 per cento. Colleghi, lo diciamo con chiarezza: la legge in discussione sulla rigenerazione urbana è fondamentale e va riscritta *(Applausi)*, perché deve servire a realizzare innovazioni nelle città, non a musealizzare

e che il Governo trovi delle risorse. Ci sono infatti poi altre questioni di fondo per finanziare la ripresa. Quando io leggo che in Europa Amazon ha 44 miliardi di entrate e paga zero euro di tasse dico che anche qualche *rapper*, invece di fare il *testimonial* di Amazon,

ci sia da lavorare anche su questi versanti, tutelando il mondo del lavoro, le aziende, le imprese, ma anche il mondo delle professioni e delle partite IVA. Questo è lo spirito con cui noi partecipiamo - senza essere subalterni a nessuno, ma consapevoli di una fase di emergenza - a questo momento che condividiamo come uno sforzo nazionale, come hanno detto i nostri colleghi che sono intervenuti nel dibattito, che hanno lavorato in Commissione, con la certezza che la svolta di Governo sia stata essenziale per fare rispettare di più l'Italia in Europa, per cominciare a rivedere i meccanismi di quel *triplete*: più vaccini,

giunge oggi al termine una vicenda legislativa che è nata in un clima economico e politico completamente diverso, sul quale varrà forse la pena di spendere qualche parola proprio per motivare il voto favorevole che ci accingiamo ad Vorrei intanto cominciare ringraziando i colleghi delle Commissioni riunite che mi hanno accompagnato nel percorso di conversione del decreto-legge; un percorso che, con un garbato eufemismo, mi permetto di definire accidentato. In un periodo in cui le regole - le cosiddette regole - che poi sono quelle che a sinistra una volta si sarebbero chiamati i rapporti di forza, si stanno sbriciolando - come da noi più volte auspicato e preconizzato - lasciatemi dedicare un commosso pensiero di solidarietà al Regolamento, che invece spero resti saldo a tutela di tutti, soprattutto a tutela di quel bene prezioso che, se purtroppo è veramente razionato dalla natura, è il nostro tempo. Tempestività non fa rima con frettolosità e nemmeno con arbitrarietà, ma scordiamoci questa esperienza. Il percorso del provvedimento nasce il 15 gennaio scorso, quando il precedente Presidente del Consiglio presentò alle Camere una relazione ai sensi della legge n. 243 del 2012, chiedendo uno scostamento di bilancio da 32 miliardi. Il presupposto dell'intervento era l'introduzione di nuove misure restrittive che erano state prese a dicembre e poi consolidate con il decreto-legge n. 2 del 2021 e con il DPCM del 14 gennaio. La finalità era quella di fornire un ulteriore sostegno alle categorie colpite dalle misure restrittive, che si riteneva sarebbero state relativamente transitorie. Sappiamo poi quali vicissitudini abbiano ritardato la spesa di quelle risorse. La crisi di Governo ha portato a emanare il decreto-legge sostegni solo il 22 marzo scorso; sappiamo anche che le misure restrittive sono proseguite e sono ancora in vigore, con diversi gradi di intensità. La Lega, scegliendo con senso di responsabilità di sostenere questo Esecutivo non di unità ma di salvezza nazionale, è riuscita imprimere a questo provvedimento la sua cifra di buon senso e di concretezza. Se da qualche mese non sentiamo più parlare di codici Ateco, è perché questo provvedimento accoglie, fra le altre, una nostra specifica richiesta più volte espressa in queste Aule *(Applausi)*. Anche l'innalzamento del tetto di fatturato da 5 a 10 milioni, pur con i limiti che l'arbitrarietà di qualsiasi soglia definita porta con sé, ha contribuito ad allargare la platea dei beneficiari e segue una nostra richiesta. Infine, a più di un anno dall'inizio della crisi e con la tempestività di analisi dei dati offerta dalla fatturazione elettronica, non aveva più senso ricorrere a un criterio di idoneità arbitrario come il calo di fatturato nel solo mese di aprile, che penalizzava ingiustamente tante attività caratterizzate da andamento stagionale. Anche il criterio di idoneità del mese di aprile, da noi sempre contestato, è stato aggiornato e migliorato nel provvedimento in esame, prendendo come riferimento il fatturato non di un mese, ma il fatturato medio mensile. Altra e non meno importante richiesta che la Lega aveva avanzato fin dal mese di novembre l'anno bianco contributivo, che nel provvedimento in esame viene rifinanziato con esonero dai contributi previdenziali minimi dei lavoratori autonomi colpiti da un calo di fatturato. Tale misura affianca quelle prese a tutela del lavoro dipendente con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. negli infiniti dettagli della misura. Siamo ormai abituati a provvedimenti di urgenza che hanno le dimensioni di una legge di bilancio. Ma, se volessimo discuterli adeguatamente, dovremmo riformare il Regolamento dando alla discussione altri tempi. L'elenco delle tante cose fatte in Parlamento, sia pure con risorse limitate per migliorare il decreto-legge, è stato fatto in discussione generale. Vorrei dire con chiarezza che credo siamo tutti consapevoli dei limiti che anche questa misura necessariamente porta con sé e siamo naturalmente grati all'opposizione che, svolgendo il suo ruolo, ci aiuta in questa importante crescita di consapevolezza. I limiti della misura derivano in primo luogo dal fatto di essere stata concepita in tempi in cui si riteneva che le misure restrittive sarebbero state più circoscritte nel tempo e dal fatto che una crisi di Governo ha ritardato l'erogazione dei fondi. Dobbiamo però contestare e distanziarci da polemiche sterili come quella che, equivocando spregiudicatamente sul criterio di idoneità definito sulla media annua del fatturato mensile, ha accusato questo Governo di voler compensare con un indennizzo irrisorio la perdita di fatturato del 2020. L'indennizzo, in effetti, andrebbe commisurato ai mesi di ulteriori clausura previsti al momento in cui lo stanziamento è stato disposto (dicembre-gennaio) e non all'anno 2020. I numeri ci dicono che con il provvedimento in discussione questo Governo ha dedicato ai contributi a fondo perduto una somma pressoché identica a quella che il precedente Governo aveva allocato in quattro decreti-legge è già in arrivo il primo provvedimento interamente concepito dal Governo in carica, il secondo decreto-legge sostegni, finanziato da uno scostamento da 40 miliardi e indirizzato al mondo dell'impresa. Questi sono i numeri di questo Governo e questo è un cambio di passo documentabile. Dopodiché, senza tema di compromettere la serenità del clima esterno e interno a quest'Aula, mi permetto di osservare quello che tutti sappiamo e che la stessa relazione sullo scostamento del 15 aprile dice con chiarezza: l'esperienza dimostra che il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena la vita sociale, economica e culturale si riavvicina alla normalità. Ecco: normalità, proporzionalità degli interventi. Se guardo in alto, oltre il velario che riporta le effigi dei padri della nostra civiltà giuridica, vedo più su affacciarsi da una nuvoletta l'inconfondibile fisionomia sorniona di Giorgio Gaber e mi immagino il suo divertimento nel constatare che oggi, oltre al culatello o alla giacca, anche certe molecole sono di destra, mentre, oltre alla mortadella o ai *jeans,* anche chiudere è di sinistra Chiedo scusa ai colleghi progressisti per lo psicoreato di utilizzo abusivo di una loro icona, ma assicuro che è stato fatto a fin di bene, per attirare la loro e la nostra attenzione su un punto. la verifica sull'efficacia e la fondatezza delle misure di intervento non farmaceutico (cioè sostanzialmente delle chiusure, per capirci), che la Lega ha chiesto e ottenuto per metà maggio, possa svolgersi in un clima sereno e nutrirsi di valutazioni basate sui fatti e sulla letteratura scientifica vera, non su quella dei *talk show*. Abbiamo visto un'altra stagione di guitti da *talk show*, quelli che difendevano l'austerità; viene da dire che in questo caso la storia si è ripetuta, prima come farsa e ora come tragedia. Il vero sostegno all'economia sarà liberarla, naturalmente laddove ci sia un fondamento scientifico per farlo; ma questo fondamento non ci sarà se il dibattito si fossilizzerà su preconcetti ideologici, quelli verso cui Gaber manifestò divertita e motivata insofferenza, e se si confonderà la scienza con lo scientismo. Ve lo dico contro il mio interesse, perché, se invece si ragiona così (confondendo scienza e scientismo), poi si finisce come a Madrid; l'aspirazione alla libertà è incomprimibile e a chi ha voluto comprimerla, quale che ne fosse il motivo, la storia ha sempre presentato un conto salato, nel migliore dei casi in termini elettorali. Guardiamo quindi al futuro con fiducia, ma soprattutto con razionalità, e intanto votiamo favorevolmente questo provvedimento.

Signora Presidente, Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, finalmente siamo qui in Aula per votare il decreto sostegni. Eravamo partiti a gennaio, con il Governo Conte due in carica, con la votazione dello scostamento di 32 miliardi di euro, che servivano per questo decreto-legge, che avrebbe dovuto essere il ristori Stavamo procedendo spediti e avevamo aperto un'autostrada davanti a noi, per far arrivare quanto prima sul territorio gli aiuti messi in campo. Poi qualcuno ha deciso che si doveva fermare in autogrill per un appuntamento, abbiamo perso tempo, cambiato autista e ora siamo qui con una nuova squadra a parlare dello stesso provvedimento. Per fortuna all'irresponsabilità e alla spregiudicatezza di qualcuno ha fatto da contraltare l'enorme responsabilità di altre forze politiche, a partire dal MoVimento 5 Stelle. Ma ci siamo; l'importante ora è che i 32 miliardi arrivino sul territorio, perché alle persone e alle aziende che sono al di fuori di questo Palazzo non interessa chi sia oggi alla guida o i problemi politici interni, ma interessa che siano aiutate e supportate. Vorrei porre l'attenzione sul fatto che questo ennesimo provvedimento economico, il dodicesimo da quando è scoppiata la pandemia, non va assolutamente visto come un intervento a sé. Esso fa parte di un percorso, integra e sviluppa quello che abbiamo chiamato il treno dei ristori; lasciamo perdere il fatto che oggi si chiamano sostegni, perché la sostanza è quella. Se andiamo a prendere il singolo intervento, come è stato detto anche in quest'Aula, è chiaro che da solo non è sufficiente; ma, se consideriamo complessivamente il cura Italia, il liquidità, il rilancio, il semplificazioni, il decreto agosto, i ristori, gli altri decreti minori, la legge di bilancio, il sostegni uno e l'imminente ci rendiamo conto che con dodici provvedimenti economici abbiamo immesso nel sistema già circa 200 miliardi. Si tratta di soldi che servono per aiutare le nostre aziende, i professionisti e i cittadini per aiutare il nostro Paese, senza tener conto dei soldi che metteremo e che arriveranno con il PNRR, che si occuperà della parte di investimenti e di rilancio dell'Italia per i prossimi sei anni.

Quando abbiamo iniziato con il primo decreto a marzo 2020, tutti speravamo che i tempi bui durassero solo pochi mesi; ma, non avendo vissuto mai situazioni di pari entità, ci siamo dovuti organizzare per fornire il supporto necessario alle imprese e alle persone che ne avevano bisogno. Così sono nati il decreto rilancio e tutti gli altri decreti. Questo, di base, è il primo vero provvedimento del Governo Draghi in cui si decide delle risorse che verranno impegnate a breve, oltre al PNRR (ma lì parliamo di investimenti a medio e lungo vogliamo, il banco di prova della tenuta di questa maggioranza, perché discutere di temi e soluzioni in una maggioranza così allargata non è facile; tantomeno è facile mettersi d'accordo quando ci sono posizioni divergenti. In alcuni casi sono stati raggiunti punti di intesta soddisfacenti per tutti, mentre in altri si è deciso di lasciar correre: vedi il superbonus, per cui, nonostante la spinta del MoVimento 5 Stelle e la volontà di intervenire sin da ora, il resto della maggioranza ha ritenuto di non voler intervenire. Pure il presidente Draghi ha detto che dobbiamo semplificare il processo e che non avevano senso i ritardi sulle misure che non avevano un impatto economicamente, ma solo in termini di snellimento del processo. In altri casi, invece, è stato concesso a qualcuno, in virtù di sbandierati accordi di Governo fatti in quest'Aula, di portare a casa una bandierina, pur sapendo che la lotta in questione era stata portata avanti anche da altri Gruppi politici. Chi sa come sono andate le cose, che siano aziende, professionisti o semplici cittadini che hanno visto nel tempo chi o quale Gruppo politico si è davvero interessato alla materia, non si farà ammaliare da un *post*, da un lancio di agenzia o da un comunicato stampa. Comunque, a noi del MoVimento 5 Stelle interessa che questo decreto-legge vada in porto, perché quando diciamo che ci interessano tutti e che nessuno deve restare indietro, per noi non è uno *slogan* ma è la ragione del nostro essere qui. non dimentichiamo mai che dietro a ogni situazione ci sono delle persone cui andare incontro. In questa dichiarazione di voto voglio parlare di due emendamenti: uno è presente nel documento che oggi verrà approvato, e l'altro è stato invece stralciato oggi, pur essendo stato approvato in Commissione. Entrambi però dimostrano quanto il MoVimento 5 Stelle tenga a supportare il nostro tessuto produttivo. Nel primo caso, con un nostro emendamento presentato a mia prima firma,

e che rischiavano di essere escluse o penalizzate anche dal meccanismo previsto dal decreto-legge sostegni, ritrovandosi in una sorta di limbo. L'esempio classico è quello delle partite IVA aperte nel 2018 che, per una serie di motivi, hanno cominciato a fatturare magari solo a partire dalla seconda metà del 2019. Prendiamo per esempio un bar, un ristorante, un negozio: dal momento della costituzione della società nel 2018, tra ricerca del locale, messa a norma, ristrutturazione e autorizzazioni, magari hanno emesso il primo scontrino solo nel 2019, di fatto restando esclusi dal decreto-legge sostegni, così come lo è stato dal decreto-legge ristori. Ora non più: con la riformulazione proposta dal MEF è stato previsto un contributo a fondo perduto di 1.000 euro, che possiamo considerare in ottica positiva un bicchiere mezzo pieno. La buona notizia è che adesso c'è un bicchiere e c'è anche un po' d'acqua dentro. Ora toccherà al Governo e alla Camera, nel prossimo decreto-legge, cercare di chiudere e completare questo ammontare di risorse che serviranno a ristorare tutti. L'altro emendamento di cui vi voglio parlare è invece quello che aveva presentato il nostro collega Turco, sulla cessione a terzi dei crediti d'imposta, (Transizione 4.0), analogamente a quello che è previsto per il superbonus 110 La norma avrebbe concesso di dare respiro alle imprese, perché avrebbe permesso loro di creare liquidità, cedendo subito quel credito di imposta che le aziende hanno "in pancia" senza attendere lunghi mesi prima di poterlo usare.

maxiemendamento su *input* della Ragioneria generale dello Stato per potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica. Tali effetti, secondo quanto riportato nel parere presentato in Commissione, potrebbero essere estremamente rilevanti, pertanto la norma è stata stralciata. Ma questo è qualcosa che come MoVimento 5 Stelle non ci andava bene, perché sebbene accada ogni tanto che in fase di conversione di un decreto-legge durante la fiducia possano essere stralciati alcuni emendamenti, non è mai accaduto che un emendamento di portata così rilevante sia stato stralciato. Quindi o la Ragioneria generale dello Stato si è sbagliata in precedenza e noi abbiamo potuto votare in Commissione, oppure si sta sbagliando adesso. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo fermamente espresso la nostra posizione di dissenso rispetto a questa posizione, in quanto un errore così corposo da parte di una struttura che deve essere di supporto al Parlamento non può succedere e non deve più succedere.

Tutte le imprese hanno infatti bisogno di questo supporto. Signor Presidente, stanno aumentando le vaccinazioni. Dobbiamo ancora stare attenti e tutti ci auguriamo che le riaperture in corso siano un segnale positivo che non venga interrotto da una recrudescenza del virus. Come MoVimento 5 Stelle ci auguriamo che i prossimi provvedimenti siano maggiormente orientati a dare una spinta all'Italia per tornare verso la regolarità, con supporti che riguardino sempre più la ripresa della normalità della vita del Paese (e Transizione 4.0 era uno di quelli). In tutto questo, il decreto sostegni, che - ripeto - fa parte di un treno partito con il Conte II e che ha effettuato numerose soste, è un altro tassello fondamentale per aiutare l'Italia. Sappiamo che non sarà l'ultimo nonostante le diverse soluzioni proposte, che spaziano in maniera ampia, come ampia è la maggioranza estremamente variegata che supporta questo Governo, e nonostante questa brutta pagina, che siamo sicuri verrà risolta a breve grazie anche alla rassicurazione del ministro Franco, posso dichiarare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. Signor Presidente, la cedibilità dei crediti non c'è, caro MoVimento 5 Stelle. Non c'è sul superbonus e nemmeno su altri *bonus*. Il decreto sostegni è quindi un sostegni bla bla, per cui voterete una fiducia bla bla. Domani inizierete un tavolo di lavoro; sempre domani voi volete fare le cose. Domani volevate abbassare le bollette della luce e del gas, abbattendo gli oneri di sistema; ma, appunto, è domani. «E se domani (e sottolineo se)», cantava Mina. Ma l'amico Licheri non è Mina, non ha la sua voce. Oggi la ristorazione piange, come piangeva ieri, stritolata dalle vostre assurde norme: siamo al 6 maggio e c'è ancora il coprifuoco alle ore è stritolata dalle banche, che vogliono umiliare le famiglie e i piccoli operatori economici; è stritolata dalle multinazionali del *delivery*, quelle multinazionali a cui non avete torto un solo capello. Le multinazionali evadono il fisco che è una bellezza, perché lo fanno a norma di legge. Ai ristoratori fate le multe, alle famiglie e agli imprenditori togliete la cessione del credito e al turismo mettete uno stupido *pass* vaccinale, per cui si deve pagare per potersi fare i tamponi e i *test* sierologici: un *pass* sulla base del reddito. Il comparto dei matrimoni aspetta un protocollo chiaro e vi domando: bisogna vincere lo scudetto per fare la festa? A proposito di feste, per le banche è sempre festa, ma per Montepaschi lo è sempre un po' di più, perché il Governo ci sta nascondendo la verità su MPS. Perché non promuovete l'azione di responsabilità contro Profumo? Gli italiani a cui date ristori e sostegni bla bla devono sapere che i bilanci di MPS sono stati truccati e che i nostri soldi sono serviti per tamponare quei giochi di prestigio. Oggi una perizia di quasi seimila pagine ha evidenziato che sui crediti deteriorati gli ex vertici della banca hanno violato le normative. Perché Draghi non parla? Perché Daniele Franco non parla? Perché il PD e il resto della maggioranza non parlano? Ci sono di mezzo i soldi degli italiani. E allora, se c'è da dire la verità, l'unico sostegno che interessa a questo Governo è il sostegno a banche e multinazionali: quello vi riesce molto bene. Complimenti! Italexit voterà no.

tutto ciò che era stato proposto da una certa parte politica e che realmente sarebbe servito al Paese è stato stralciato. Così sono stati tolti il superbonus per le imprese, che consentiva la cedibilità dei crediti di imposta, e altre misure. Tutto ciò che era cedibile e che dava ossigeno alle imprese è stato tolto; è stata tolta l'impignorabilità del reddito di cittadinanza, mentre sono stati dati segnali chiari, come, ad esempio, quello del condono, che è devastante: è il segnale che i furbi hanno dei vantaggi. Ho sentito alcuni oggi dire che quello che è accaduto è inaccettabile, però poi lo accettano; per L'Alternativa C'è, invece, ciò che è inaccettabile resta inaccettabile. Voteremo quindi contro questo provvedimento. Signora Presidente, onorevoli senatori, chiedo la parola per annunciare e motivare il mio voto in dissenso sul decreto sostegni, che tra tante misure indispensabili per accompagnare imprese e cittadini in questo difficile momento, ne contiene una, quella relativa al condono fiscale, inaccettabile per tutti i contribuenti onesti e pesantemente bocciata, oltre che da milioni di cittadini e dalle forze sindacali, da alcune delle massime autorità di questo Paese: Corte dei conti, Banca d'Italia, per non parlare dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Ho sostenuto la costituzione di questo Governo per affrontare i tre punti necessari per superare l'emergenza pandemica indicati dal presidente della Repubblica Mattarella e nel discorso programmatico del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi in quest'Aula del 17 febbraio scorso: la lotta all'evasione...

La lotta all'evasione, che solamente nell'ultimo anno è ammontata a 107,2 miliardi, era uno degli impegni prioritari. Mai perciò mi sarei aspettato da questo Governo la proposta del solito condono in regalo agli evasori, che tra l'altro per la prima volta nella storia ha anche un costo rilevante per le casse pubbliche: almeno 700 milioni di euro; oltre al danno, dunque, anche la beffa. Ci dite, voi rappresentanti del Governo, che questo condono andrebbe fatto per sgravare il magazzino della riscossione da cartelle non più riscuotibili. Sapete bene che questo non è vero, perché secondo i dati della stessa Agenzia delle entrate le cartelle effettivamente non più riscuotibili, perché relative a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, sono il 40 mentre il resto fa capo a contribuenti perfettamente in grado di versare il dovuto. Siamo di fronte quindi al solito gioco: i partiti si ingraziano gli evasori sperando di incamerarne i voti. Vince così ancora una volta il partito trasversale dell'evasione fiscale evidentemente fortissimo anche in questo Parlamento. Ma attenzione: vincete lanciando un messaggio devastante di ingiustizia al Paese, dicendo ai contribuenti che evadere le tasse conviene, tanto prima o poi arriverà il solito condono. Vincete lasciando il peso del sostegno delle casse pubbliche e del *welfare*, che gli evasori utilizzano a man bassa...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

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Colleghi al fine di non creare confusione, vi avverto che ci sono state molteplici richieste di anticipo del voto. In base a quello che mi è stato indicato dai singoli Gruppi, io non ho opposto eccezioni. Quindi, partendo dal Governo, ognuno di voi poi potrà chiedere al proprio Capogruppo.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: